L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Segretario. Ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulterà eletto il senatore appartenente al Gruppo Misto che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa. La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Dopo la chiama le urne resteranno aperte fino alle ore 12. Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

Stefani

*(Applausi)*. Oggi assistete, in realtà, a una seduta particolare. Come vedete, ci sono due urne davanti alla Presidenza, perché stiamo eleggendo un senatore Segretario. Le urne sono aperte la Presidenza è in attesa che qualche senatore che ancora non lo ha fatto venga a votare. L'Aula è vuota perché, in contemporanea, i senatori sono impegnati alla Camera dei deputati per eleggere i giudici della Corte costituzionale. Siete quindi entrati in un momento speciale. **Ripresa

appena visto come si svolge una votazione in urna. Il senatore viene chiamato, entra in cabina e scrive la propria preferenza. Vi è un'urna all'uscita, dove viene inserita

11)** Colleghi, riprendiamo i lavori dell'Assemblea, intesi come trattazione dei punti all'ordine del giorno.

per l'anno finanziario 2023) e 4 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2024).

e la sua idea dei detenuti che soffocano nelle automobili, di cui abbiamo avuto tutti contezza nei giorni scorsi. In quell'articolo, di questi sedicenti comunisti proletari, si citava, tra i tanti che hanno criticato le parole del sottosegretario Delmastro, il collega Verini.

del Governo nei confronti di un esponente dell'opposizione. Noi ci tenevamo a sottolineare questa cosa, che per noi è inaccettabile, e chiediamo al ministro Nordio se condivida questo modo di comportarsi del sottosegretario Delmastro nei confronti di esponenti dell'opposizione.

I "proletari estremisti" invocano violenza e pena di morte contro di me, reo di difendere leggi e divise, citando Verini come ispirazione. Non ci faremo intimidire. saremo sempre con lo Stato, le Forze dell'ordine e la giustizia contro l'odio». È oggettivo che questi sciagurati proletari comunisti abbiano citato il senatore Verini, ma Delmastro non ha detto nulla contro il senatore Verini. Loro lo hanno citato e mi dispiace per il senatore Verini, che penso non si riconosca nelle posizioni espresse; semmai dunque il dispiacere è nei confronti del senatore Verini. Il sottosegretario Delmastro ha parlato

ma è oggettivo che questi sciagurati comunisti proletari hanno lanciato minacce di morte al sottosegretario Delmastro e che hanno citato il senatore Verini. Mi dispiace davvero, sinceramente, per il senatore Verini, ma mi dispiace anche per il sottosegretario Delmastro, minacciato di morte.

Signor Presidente, siamo qui perché, come ogni anno, l'Assemblea del Senato si trova a esaminare gli atti relativi al bilancio interno di questa istituzione. Questa volta si tratta del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2023 e del progetto di bilancio riferito all'anno 2024, che il Consiglio di Presidenza ha deliberato nella riunione di ieri 27 novembre. Limitandomi a un esame essenziale di questi due documenti contabili, iniziando dal bilancio relativo all'anno 2024, osservo, innanzitutto, come la spesa complessiva finale sia rimasta invariata rispetto al bilancio inerente allo scorso anno, nonostante l'attuale dato inflattivo. Tra l'altro, le entrate del Senato evidenziano che la dotazione finanziaria è rimasta invariata dal 2012, nella misura di circa 505 milioni di euro. Per conseguenza, rispetto alla dotazione richiesta nel 2011, pari ad euro 526.960.500 si registra una riduzione annua di 21,6 milioni di euro. Tenendo conto che l'importo della dotazione rimarrà invariato anche nell'esercizio 2024, così come si può evincere dal bilancio di previsione per l'esercizio in corso, la riduzione cumulata dall'inizio della scorsa legislatura risulta pari addirittura a 200,8 milioni di euro. La costante riduzione della spesa negli ultimi anni si è dunque accompagnata ad di euro. La costante riduzione della spesa negli ultimi anni si è dunque accompagnata ad una sostanziale stabilità della principale entrata del Senato, con l'assestamento di quest'ultima su un livello significativamente più basso rispetto agli anni antecedenti alla crisi del 2011. Si registra, per quanto riguarda la spesa di funzionamento, una riduzione del 1,17 per cento rispetto al 2023 e un leggero aumento, pari all'1,42 per cento, della spesa di natura previdenziale. Occorre evidenziare, inoltre, la circostanza che nello scorso anno finanziario la spesa corrente nel suo complesso è aumentata solo dello 0,1 per cento, restando pertanto nel suo complesso invariata rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione di un'ottima gestione delle risorse pubbliche in periodi di significativa inflazione quale quello attuale. Viceversa, risulta in diminuzione la spesa in conto capitale che, tra il 2023 e il 2024, passa da 7,13 milioni di euro a 6,255 milioni. La spesa in conto capitale, che costituisce l'aggregato meno rilevante in termini assoluti tra quelli precedentemente precedentemente citati, comprende le spese per l'acquisto di beni mobili inventariati, le spese di manutenzione straordinaria, nonché quelle di acquisto e conservazione del patrimonio della biblioteca e dell'archivio storico. A fronte di un così marcato di un così marcato contenimento della spesa, come quello registrato a partire dal 2012, la sfida, naturalmente, è stata ed è tuttora quella di rendere compatibili i risultati finanziari conseguiti: essi testimoniano la partecipazione del Senato allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica, compiuto negli ultimi anni, con il mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dei servizi erogati, tanto più in un contesto che ha visto, almeno negli ultimi anni, una costante riduzione del personale di ruolo dell'Amministrazione.

*senatore Questore*. Signor Presidente, senatori, a nome del Collegio dei Questori, quindi anche dei colleghi senatori Antonio De Poli e Marco Meloni, presento all'Assemblea il bilancio di previsione per il 2024 e il rendiconto di gestione per il 2023. Sono veramente felice e soddisfatto di poter annunciare che, anche quest'anno, il bilancio consuntivo del Senato conferma l'efficacia delle politiche di contenimento dei costi e l'affidabilità delle previsioni di spesa. Nel 2024 i risparmi ammontano a 10 milioni di euro, con una riduzione totale di 20 milioni di euro dall'inizio di questa legislatura. Mi preme richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un dato virtuoso: dal 2012 (ormai sono trascorsi dodici anni) le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il funzionamento del Senato sono diminuite di 429 milioni di euro. In questi anni abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione strutturale: pur realizzando risparmi, abbiamo continuato ad investire per rafforzare la nostra istituzione, che rappresenta il tempio delle regole e anche della democrazia per tutti i cittadini. Ci siamo riusciti ottimizzando le risorse, superando la logica dei tagli puri, spesso mai accompagnata da una strategia o da una visione più ampia. Se oggi possiamo presentare un bilancio virtuoso del Senato, significa che abbiamo lavorato tutti insieme, senza posizioni ideologiche e senza nessuna strumentalizzazione, per perfezionare il funzionamento di questa importantissima istituzione. Questo risultato straordinario evidenzia la capacità dell'Assemblea e della sua macchina amministrativa di saper rispondere alle difficoltà dei cittadini che, in un periodo segnato da questi enormi sacrifici, meritano sempre più rigore e buon senso nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La scia virtuosa di questo cammino verso un progressivo e anche costante calo dei costi è stata resa possibile grazie a un processo di revisione sistematica, strutturale e soprattutto funzionale di ogni capitolo di spesa. Queste procedure di efficientamento ci hanno permesso di aumentare la qualità e il numero dei servizi a disposizione sia dei singoli senatori sia degli organi, come le Commissioni e i Gruppi parlamentari. Nel corso di quest'anno le spese di funzionamento sono state ridotte di quasi 4 milioni di euro e le spese in conto capitale sono state ridotte di quasi un milione di euro con una contrazione dell'11,5 per cento. Considerato anche l'aumento dei prezzi degli ultimi due anni, con l'inflazione che nel 2022

Infatti, se consideriamo l'effetto dell'inflazione, il valore reale della dotazione del Senato dal 2011 ad oggi è stata ridotta di circa 136,4 milioni di euro; la dotazione rivalutata si aggirerebbe attorno ai 641,4 milioni di euro. Questi risultati sono il frutto di diverse ma soprattutto vorrei sottolineare che c'è stata la riduzione annuale della dotazione per 21,6 milioni di euro; ci sono stati risparmi legati a riforme previdenziali e anche a misure di solidarietà per ex senatori ed ex dipendenti, con un risparmio di 27,1 milioni di euro, oltre ai 17 milioni del periodo che va dal 2014 al 2016. Ci sono state efficienze anche derivanti dai processi di razionalizzazione della spesa, con risparmi che sono stimati dai 9 ai 16 milioni di euro dal 2016 al 2024. Questa costante riduzione, e anche un'oculata ottimizzazione delle spese, hanno reso quindi il Senato un modello virtuoso per altre amministrazioni dello Stato. Rigore, trasparenza e anche un continuo processo di riorganizzazione delle voci di bilancio strutturali e funzionali hanno permesso a questa istituzione di adempiere pienamente ai suoi compiti costituzionali; un ruolo che spetta ai parlamentari, a tutti i dipendenti e ai funzionari impegnati ogni giorno a rappresentare la sovranità popolare. In quest'ottica, il Collegio dei Questori ha il dovere di garantire anche il miglior funzionamento dell'istituzione, attraverso una gestione prudente e trasparente dei processi gestionali, senza mai compromettere la qualità del servizio offerto al Paese. Per quanto riguarda gli impegni presi con gli ordini del giorno approvati nella precedente sessione di bilancio interno, il Collegio dei Questori ha completato l'istruttoria sulla disciplina del trattamento economico dei collaboratori dei senatori in relazione all'attività svolta. Annunciamo oggi una nuova delibera, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, per disciplinare il rapporto di lavoro tra senatore e collaboratore e il conseguente trattamento economico in relazione all'attività svolta. Permettetemi di dire che questo è un primo passo fondamentale per restituire dignità sociale ai collaboratori parlamentari, non solo tutelando i loro diritti,

lavoro dall'intero Consiglio di Presidenza, affiancato in ogni momento dalla grande professionalità di tutta l'Amministrazione del Senato, che ha consentito di dare attuazione ai diversi impegni assunti con gli altri ordini del giorno trattati nella precedente sessione di bilancio interno.

il Senato. Sempre in attuazione degli ordini del giorno, abbiamo previsto l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche idonee a favorire sia in Commissione, che in Assemblea un miglior coordinamento

Tra questi, ricordo la possibilità, anche in situazioni di particolare rilevanza istituzionale e culturale, di fornire direttamente un servizio di interpretariato e traduzione di lingua dei segni italiana all'interno delle trasmissioni in *streaming* della WebTv del Senato. Abbiamo anche raccolto l'invito, sempre da parte del MoVimento 5 Stelle, a una migliore tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nelle singole commesse e nei contratti di appalto di servizi e forniture stipulati dal Senato.

Ringrazio il presidente Ignazio La Russa per il modo in cui, in questi due anni, ha presieduto l'Assemblea, tutelando tutte le forze politiche senza alcuna distinzione. Non posso fare a meno di esprimere infinita gratitudine a tutta l'Amministrazione del Senato, cuore e motore di questa grandissima istituzione, a partire dal segretario generale, dottor Federico Silvio Toniato, e ai quattro vice segretari generali *(Applausi)*, dottor Alfonso Sandomenico, dottor Edoardo Sassoli, dottor Alessandro Goracci e dottoressa Grazia Maniscalco, per l'impegno incessante e fondamentale che dedicano ogni giorno per l'ottimo funzionamento del Senato. Un affettuoso ringraziamento a tutti i direttori dei Servizi, *in primis* al direttore del polo medico sanitario, dottor Federico Marini, e a tutti i dipendenti *(Applausi)*, lavoro essenziale, ma anche silenzioso, rendono possibile la nostra attività, dai collaboratori dei senatori e dal personale dei Gruppi parlamentari a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri, ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale di Roma Capitale, che ogni giorno garantiscono la sicurezza di questi Palazzi ricchi di storia, di arte e di cultura. Desidero altresì salutare i senatori presenti oggi al dibattito e, in particolare, ringraziare quanti interverranno anche per arricchirlo con preziosi suggerimenti. Il Senato lavora ogni giorno per riconnettere quei tanti nostri concittadini che avvertono le istituzioni lontane ed estranee alla loro vita e per intendere la politica come servizio al bene comune, che è patrimonio di ognuno di noi. La democrazia non è una conquista definitiva, ma va realizzata continuamente, individuando le formule più adeguate al mutamento dei tempi. Il fatto che questa Assemblea individui le soluzioni più appropriate ai bisogni attuali rappresenta proprio il principio di una democrazia viva e dinamica che si nutre chiaramente del contributo attivo dei cittadini e dei rappresentanti eletti all'interno delle istituzioni. In tal senso, dimostriamo anche quest'anno di saper essere flessibili e di saper rispondere ai nuovi bisogni, alle sfide del presente e del futuro.

senatore Questore Nastri anche per averci ricordato che il bilancio non è una semplice, seppur importantissima, questione contabile, ma stiamo discutendo del funzionamento di uno dei principali luoghi,

ha evidenziato il collega Nastri qualche minuto fa, che in due anni abbiamo risparmiato 20 milioni; 429 milioni dal

È importante capire quello che abbiamo fatto in questi anni; non abbiamo tagliato, ma razionalizzato, controllato, verificato, messo insieme tutte le varie voci di bilancio, facendo nuovi lavori e introducendo una serie di innovazioni con innovazioni con attenzione, come se fossero questioni di casa nostra. Credo che questo sia l'aspetto per cui ancora oggi stiamo avendo un bilancio positivo *(Applausi)* e con risparmi, ma senza particolari tagli.

di cui in questi ultimi tempi si sta parlando in moltissimi settori, per una maggiore efficienza nel supporto delle nostre attività parlamentari e, in modo particolare, per la resocontazione in Assemblea e nelle Commissioni, per la classificazione degli atti parlamentari e per l'analisi di tutti i testi legislativi. Credo che questo sia un aspetto virtuoso e importante. Uno degli atti altrettanto positivi riguarda il fatto che non a caso noi paghiamo i nostri

più importante, ma altrettanto difficile. Ricordo l'accessibilità ad esempio, alla Nassirya, l'accessibilità all'ingresso di palazzo Carpegna, la nuova riorganizzazione dell'ingresso tra Carpegna e Madama, e moltissimi altri interventi. Questo significa avere attenzione verso tutti e credo che un'istituzione come il Senato debba sempre averla come priorità.

menzionare tutte le auto che sono elettriche o ibride, i contenitori della raccolta differenziata e tutta una serie di altri interventi che abbiamo fatto. Ricordo che il rapporto tra la spesa del Senato e la spesa del bilancio dello Stato è molto importante per quello che riguarda il Senato. Pensate che per 100 euro dello Stato, noi abbiamo quattro centesimi: anche quest'anno abbiamo diminuito ulteriormente Il contenimento della spesa per la retribuzione del personale è del 20 per cento e lo stesso riguarda l'indennità parlamentare. Credo che questo sia uno degli aspetti altrettanto importanti.

Ricordo tutti i servizi tecnici, come dicevo prima, dalle barriere architettoniche a tutto il resto che si sta facendo per dare un miglior funzionamento delle nostre attività. Ricordo, non per ultimo, che all'interno di ognuno dei

il dottor Federico Marini, che è sempre attento a ognuno dei nostri problemi, che ci possono essere normalmente all'interno della vita del Palazzo e non solo. Vorrei ringraziare tutte le Forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco, e i Vigili urbani che

dell'attenzione che vorrete dedicarmi in pochi secondi, perché vorrei semplicemente associarmi a tutti i ringraziamenti, che sono piuttosto lunghi, ma che faccio veramente di cuore, a tutte le persone

i numeri fondamentali sono stati descritti molto bene dai colleghi, che ringrazio perché lavoriamo bene insieme, e non è una cosa scontata. Ringrazio anche tutte le colleghe e i colleghi che ci consentono di recepire le istanze e i tanti Grazie a tutti finalmente si introduce la disciplina dei contratti dei collaboratori, un passo in avanti molto importante. Così come è molto importante il fatto che il Consiglio di Presidenza, nell'approvare ieri la delibera che aveva - appunto - questo - questo punto come oggetto, abbia disciplinato in via sperimentale, in maniera più semplice e flessibile, questo rapporto, per pochi mesi; perché entro sei mesi noi vorremmo - come descrive molto bene e come ci richiama a fare la delibera - giungere a una definizione più complessiva e completa dei compiti e dei diritti di tutte le persone che collaborano con noi, con le senatrici e i senatori di questa Assemblea. Ciò al fine di stabilire il contratto collettivo nazionale di riferimento, il il numero minimo di ore, i compensi minimi, insomma tutto ciò che costruisce, attorno al lavoro dei collaboratori dei parlamentari, un *set* di diritti che renda pienamente merito ad una professionalità assai preziosa, se non decisiva per il lavoro di tutti noi.

ringraziando tutte le persone che lavorano in Senato per la loro collaborazione preziosa, per il lavoro durissimo e per l'attaccamento alle istituzioni. *(Applausi)*. Faccio naturalmente il nome del segretario generale Federico Toniato e dei suoi vice Grazie a tutti tutti, fino all'ultimo assunto in ordine di tempo, perché senza la vostra collaborazione il nostro lavoro sarebbe impossibile. Nel ringraziare i colleghi, annuncio il mio voto favorevole. Approfitto di questa occasione per rubare all'Assemblea soltanto due o tre minuti, per dire che le notizie che il collega Nastri ci ha dato sui nostri collaboratori parlamentari sono incoraggianti. Credo che noi dobbiamo restituire il senso dell'importanza di questo luogo. Non concentrarci soltanto il Parlamento costi, ma soprattutto su quanto il Parlamento produca, cioè su quali siano la sua efficienza, la sua produttività, la qualità del suo lavoro.

degli Stati Uniti, dove ci sono soltanto 100 senatori. Noi siamo reduci da quella che io considero una sciagurata riduzione del numero dei parlamentari, perché si diceva che 315 senatori erano troppi e che 200 andavano bene. I senatori degli Stati Uniti sono 100 e hanno sono 100 e hanno una cosa che si chiama *Senators' Official Personnel and Office Expense Account*, che sarebbero le spese per l'esecuzione del mandato. Ora, le spese per l'esecuzione del mandato del nostro bilancio del Senato ammontano in tutto a 10,5 milioni per tutti noi. Quanto prende per le spese per l'esecuzione del mandato un senatore degli Stati Uniti? Una media di 3.738.775 dollari a testa. La somma totale per le spese di esecuzione del mandato degli Stati Uniti è di 449 milioni di dollari: le spese di tutto il Senato della Repubblica sono 575 milioni di euro. Il Senato degli Stati Uniti spende, solo per le spese di esecuzione del mandato, quasi quanto quasi quanto spendiamo noi tutti, avendo il doppio dei senatori. E ricordate anche che negli Stati Uniti ci sono i senati statali, quindi i senatori federali hanno delle competenze che riguardano soltanto alcune questioni, mentre noi ci occupiamo di tutto. Voglio darvi un'idea ancora più approfondita, poi davvero mi fermo. Per *Administrative and Clerical Assistance Allowance*, cioè per i collaboratori veri e propri, i senatori degli Stati Uniti hanno una somma che viene stabilita sulla base della popolazione dello Stato e che parte da 2,798 milioni di dollari, se rappresentano uno Stato che ha meno di 5 milioni di abitanti (quindi, i senatori eletti in Lombardia che rappresentano 10 milioni di abitanti, dovrebbero prendere il doppio in linea di massima e invece no), mentre la somma massima è di quasi 4,5 milioni. Poi hanno diritto a 508.000 dollari a testa per i loro uffici legislativi, mentre ci sono altre spese che sono per i viaggi, eccetera.

È chiaro che ci occupiamo dell'universo mondo, ciascuno di noi e nelle varie Commissioni, e sappiamo che tutto lo scibile umano arriva sui nostri tavoli. Auspico che un giorno torneremo finalmente a dare dignità al lavoro che si fa qui, che è un lavoro importante, perché poi noi incidiamo sulla vita delle persone. Una legge scritta male è una legge che produce effetti nel mondo; dunque, dare gli strumenti alla politica per poter poter consegnare un prodotto finale, cioè leggi fatte in modo corretto, e ovviamente assoggettarsi anche a una valutazione severa sulla propria efficienza, credo che sia molto importante. Ripeto: non è una questione di *status* del Parlamento, dotare il nostro Paese e la nostra Repubblica di strumenti funzionanti, perché poi le cose che facciamo - come dicevo - incidono sulla vita dei cittadini. Quindi, voteremo sicuramente a favore, ma non abbiamo paura di affrontare a viso aperto il tema della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia della politica, perché - non bisogna vergognarsene - questo è il luogo della massima rappresentanza democratica del Paese ed è anche il luogo dove si prendono decisioni che toccano la vita di tutti i nostri concittadini.

ringrazio i nostri Questori. L'esame dei documenti contabili interni del Senato effettivamente consolida due anni di legislatura successiva alla riforma costituzionale, la quale ha portato a 200 il numero dei senatori. Di conseguenza, il rendiconto e il bilancio che ci deposita il Collegio dei senatori Questori segnano numeri certamente razionali e funzionali rispetto al nuovo ruolo della istituzione Senato. È un bilancio saldo, assolutamente in linea con quello dell'esercizio precedente, che fotografa l'attenzione dei Questori e, ovviamente, di tutto il Consiglio di Presidenza alla dinamica della spesa. Sono due anni che hanno segnato anche il passaggio di consegne ai vertici dell'Amministrazione, per cui ci sentiamo di rinnovare il nostro omaggio alla dottoressa Elisabetta Serafin, rilevando che ha lasciato in ottime mani la guida dell'Amministrazione al dottor Federico Silvio Toniato, Toniato, che ovviamente ringraziamo; e insieme al Segretario Generale ringraziamo tutti i vertici dell'Amministrazione, a partire dai Vice Segretari Generali a tutto il personale, per la dedizione e professionalità con cui davvero lavorano ogni giorno. Questa è un'Amministrazione davvero autorevole, che nel frattempo ha riempito molti degli spazi in organico che necessitavano di forze nuove e sicuramente di nuove competenze.

Anche in questo senso consentitemi di ringraziare tutto il personale dei Gruppi parlamentari, la cui disponibilità e preparazione davvero ci aiuta ad adempiere al meglio il nostro ruolo di senatori. Ringraziamo anche tutte le Forze dell'ordine che dignitosamente espletano il loro servizio. Un ringraziamento va signore delle pulizie e a tutto il personale delle pulizie, che pure ci aiuta nel suo contesto. Abbiamo apprezzato anche che il bilancio abbia riservato impegni di spesa i quali, sostenendo l'attività parlamentare, devono poter disporre di risorse adeguate al proprio complesso e delicato compito istituzionale.

per la sua guida autorevole, ma soprattutto per la sua disponibilità. A lui, a nome di tutti i senatori di Forza Italia, va il nostro grazie per essere sempre disponibile, sempre attento a mantenere

i dipendenti, i collaboratori, la macchina amministrativa del Senato della Repubblica e, in particolare, il Servizio dell'Assemblea, che ci supporta e, come dico sempre, sopporta in quest'Aula. *(Applausi)*. Il mio è quindi un ringraziamento sentito a tutti i dipendenti del Senato. Un ringraziamento personale va anche ai membri del Consiglio di Presidenza del MoVimento 5 Stelle, il senatore Croatti, la senatrice Castellone e il senatore Lorefice, e un ringraziamento particolare va ai senatori Questori, i senatori Nastri, De Poli e Meloni, per il lavoro svolto e anche per aver accolto molte delle proposte collaborative che i nostri membri del Consiglio di Presidenza hanno voluto portare portare alla loro attenzione nella redazione del consuntivo e del preventivo per le spese di funzionamento del Senato della Repubblica. Ci sono alcuni elementi qualificanti

riguarda il tema del risparmio, è evidente che in questi anni è stata fatta un'operazione, legata anche, ovviamente, al taglio del numero dei parlamentari, di riduzione dei costi dell'Amministrazione, che in percentuale non sembra così elevato, ma che in realtà deve considerare il fatto che, in una situazione di grande inflazione, riuscire a ridurre il costo della macchina nel suo complesso richiede uno sforzo doppio. Ma il plauso che deve essere rivolto

nessuno può pensare che la democrazia non abbia un costo e che la macchina amministrativa che garantisce l'esercizio della democrazia non abbia un costo.

pensare di intervenire sulla dignità del lavoro dei collaboratori parlamentari ha un costo per l'Amministrazione. Fare i concorsi e fare assunzioni ha un costo per l'Amministrazione. Questi non sono sprechi, non sono privilegi, sono i costi legittimi dell'attività politica e dell'alta attività istituzionale della Camera alta della nostra Repubblica. Altra Altra cosa è comprare libri o cose peggiori con i fondi dei Gruppi, cosa che, purtroppo, la politica in questi anni ha portato all'attenzione delle cronache in modo sempre evidente. Una cosa è dire che la democrazia ha un costo e che questo deve essere sostenuto. Altra cosa è che bisogna sostenere un costo

di sostenere dei costi, per l'esercizio del proprio mandato, superiori a quelli dei senatori italiani. Da parte nostra, dunque, ci sarà sempre un supporto a tutti gli investimenti necessari al funzionamento della democrazia e al funzionamento delle amministrazioni che reggono la democrazia, ma certamente non saremo mai dalla parte degli sprechi

quindi ai consiglieri, agli assistenti, a tutto il personale che lavora, che ci dà una mano e che ha reso questa struttura quella che abbiamo conosciuta: una struttura sempre funzionale e precisa. in particolare il nostro segretario generale, il dottor Toniato, che ha saputo dare continuità rispetto alla

per l'attenzione che hanno avuto, non solo nel tenere il bilancio sul controllo dei conti e nella gestione del risparmio, ma anche perché sono riusciti a venire incontro a quelle che sono le esigenze dei Gruppi. Ovviamente i Gruppi, per poter far politica, hanno bisogno di disporre degli strumenti necessari. Quindi, un particolare ringraziamento a loro, perché avere senatori Questori con questa attenzione e con questa dedizione indubbiamente aiuta la politica a crescere.

Stiamo attenti, però, perché, se la politica vuole tornare ad essere protagonista, come in quest'Aula tutti quanti richiamiamo spesso, deve cercare sì di adottare delle politiche giuste ed equilibrate anche sui costi della politica, ma non autolesioniste.

mi consentiranno, il segretario generale Toniato ed i Vice Segretari Generali, di non fermarmi a chiedere loro di ringraziare l'insieme del personale che lavora nella nostra struttura, ma di provare a ringraziarlo direttamente.

Non è solo nel momento in cui ragioniamo del bilancio, infatti, che dobbiamo ricordarci delle persone che sono intorno a noi, anche se ovviamente ragionare del bilancio è il momento che permette di fare dei ragionamenti. Tra questi, vi è sicuramente l'apprezzamento per un'Amministrazione che ha saputo gestire le scelte che le erano attribuite, sia in termini di efficienza sia in termini di andamento della spesa. Io credo che questo sia il primo giudizio positivo che va dato. si evince dal fatto che anche come partito non abbiamo presentato ordini del giorno in questa occasione, nel senso che abbiamo colto il fatto che i suggerimenti che erano stati dati sono stati assunti e tradotti dal Collegio dei senatori Questori e dall'Amministrazione in scelte concrete.

frutto di un lavoro fatto dai senatori Questori, ma fatto dalla sollecitudine dell'Amministrazione, è quello di guardare al lavoro all'interno della struttura del Senato secondo il principio che una delle ragioni per cui il lavoro sia buono è che le condizioni in cui lo si esercita siano positive. È quindi giusta l'attenzione che è stata messa al tema del rinnovo degli appalti e alle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, che non sono altro dai lavoratori e delle lavoratrici direttamente dipendenti dal Senato o da coloro che dipendono dai parlamentari nella forma degli assistenti parlamentari. Era un pezzo che mancava nel ragionamento del personale e dell'attenzione a questo tema. Il fatto che ci si avvii al regolamento e alla definizione non va interpretato solo solo come una modalità per dare a quelle singole persone un contratto e ai senatori e alle senatrici delle condizioni migliori per avere dei contratti regolari. Va considerato che dare dignità al lavoro, mettere le persone nelle condizioni di lavorare positivamente, di essere visibili e riconosciute è una condizione di efficienza per tutti noi, ma è soprattutto utile all'istituzione per dare il buon esempio, perché non è mai raccomandabile che da un'istituzione del Paese venga il segnale che si è disattenti al lavoro, alle condizioni, alla contrattualizzazione, alla condizione di previdenza. Ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma molto viene guardato da questo punto di vista. Siccome io sono tra chi è convinto che fare politica, poter governare un Paese, esercitare la democrazia abbia dei costi e delle responsabilità, ritengo che sulle responsabilità bisogna soffermarsi perché la demagogia della politica come pura gratuità non ha mai funzionato. Quello che si può e si deve pretendere dalla politica è una buona amministrazione, una ragionevolezza dei suoi comportamenti, ma soprattutto la responsabilità che quelle risorse non determinino nessuna distorsione, nessun peggioramento delle condizioni di nessuno. È in ragione di tutto ciò che

del Senato, a tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano in Senato per conto di altre aziende e appalti, il nostro ringraziamento e il nostro riconoscimento dell'importanza anche per noi del lavoro che quotidianamente svolgono.

Signora Presidente, desidero esprimere le mie congratulazioni al senatore Questore anziano Gaetano Nastri e agli altri colleghi Questori De Poli e Meloni del Collegio dei Questori, che ha trovato ampio consenso, come confermato dall'approvazione unanime del rendiconto e del bilancio di previsione avvenuta ieri,

Ritengo che dagli elementi illustrati nella relazione emergano aspetti di grande valore e oggettiva positività che tutti noi possiamo e dobbiamo riconoscere. Mi riferisco, in particolare, all'impegno per la razionalizzazione delle spese: un processo che implica non tagli indiscriminati, - piuttosto - un'ottimizzazione delle risorse pubbliche, senza mai compromettere la qualità del servizio offerto alla Nazione.

Le cifre che abbiamo ascoltato poco fa sono davvero importanti e confermano la scia virtuosa nella gestione dei conti di questa Assemblea: 10 milioni di euro di risparmi nel 2024, 20 milioni di euro dall'inizio di questa legislatura e, dal 2012, un beneficio complessivo di 429 milioni di euro per le casse dello Stato. In questi anni abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione strutturale. Pur realizzando risparmi, abbiamo continuato a investire per rafforzare la nostra istituzione, che rappresenta il tempio delle regole e della democrazia per tutti i cittadini. Questo percorso virtuoso è stato reso possibile grazie a un'opera di contenimento della spesa e a un costante processo di revisione sistematica, strutturale e funzionale delle voci di bilancio. Nel corso di quest'anno il Senato ha ridotto la spesa di quasi 4 milioni di euro, con una diminuzione delle spese in conto capitale di circa un milione di euro. Questi risultati sono ancora più rilevanti se si considerano le alte percentuali dell'inflazione degli ultimi due anni. Cari colleghi, voglio evidenziare questi numeri perché è vero che la democrazia ha un costo se si vogliono istituzioni in grado di svolgere il loro compito in modo efficiente, ma è altrettanto vero che tale costo deve essere giustificato eticamente, soprattutto quando i cittadini e le loro famiglie sono chiamati a fare sacrifici. Sono convinto che stiamo seguendo la direzione giusta, come dimostrano anche le risposte che il Senato ci offre oggi. Vorrei sottolineare, poi, la puntualità del Senato nei pagamenti ai fornitori. Entro trenta giorni vengono estinte le fatture, un aspetto - questo - che dovrebbe essere di esempio per tutte le altre istituzioni ed enti che, purtroppo, non riescono a offrire sempre lo stesso livello di efficienza, con gravi difficoltà per le imprese e i cittadini in generale. Gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno nella precedente sessione sono stati mantenuti: uno su tutti, la disciplina che regola il il rapporto e il trattamento economico dei collaboratori dei senatori in relazione all'attività svolta. Ricordo che sono stati raggiunti altri obiettivi qualitativi, come gli impegni di abbattimento delle barriere architettoniche e di uso consapevole delle risorse energetiche. Sono stati implementati (e continueranno ad esserlo), senza variazione di costi, i servizi offerti per la sicurezza mediante interventi informatici. Concludo preannunciando il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e ringraziando sentitamente il presidente La Russa tutta l'Amministrazione del Senato, a cominciare dal nostro segretario generale, dottor Federico Toniato che in questi mesi ha dato già un'impronta importante in termini di capacità e senso dell'equilibrio, *ad maiorem Dei gloriam*, di questa alta istituzione. Permettetemi di estendere un sincero ringraziamento - come hanno già fatto i colleghi veramente a tutti i dipendenti del Senato, che rappresentano il nostro capitale umano e che operano per lo Stato e per gli italiani, rappresentando per tutti noi un supporto insostituibile nell'attuazione delle nostre attività istituzionali.

nuova finestra"). Salutiamo gli studenti e le studentesse del liceo scientifico «Pier Paolo Pasolini» di Potenza, che assistono ai nostri lavori. Diamo loro il benvenuto.

Presidente, ringrazio il sottosegretario Albano e tutti i colleghi. Ho l'onore e l'onere, in qualità di relatrice, di fare il punto e di tirare le fila rispetto al lavoro che abbiamo svolto in 5a Commissione bilancio,

del 19 ottobre 2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, così come approvato in seno al lavoro del Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso,

tassello prodromico alla manovra di bilancio vera e propria (un collegato) e si compone di undici articoli che contengono importanti interventi in materia di investimenti e di lavoro, alcune disposizioni fiscali e disposizioni in materia di enti territoriali. Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, dai commi 1 a 5 si prevedono diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti, relative rispettivamente alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale, al rifinanziamento del Fondo unico per gli investimenti ANAS. Il comma 6 reca invece delle disposizioni finanziarie. L'articolo 1, al comma 5-*bis*, incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentari. L'articolo 1, comma 5-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 1, 6-*octies*, introdotto durante l'esame referente, è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu, al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle Regioni dell'Emilia Romagna, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto che hanno subito dei danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie del granchio blu. L'articolo 1-*bis*, comma 1, introdotto nel corso dell'esame sempre in sede referente, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo

2, introdotto in sede referente, specifica che i contratti assicurativi - stipulati obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia - prevedono la copertura dei danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, per i beni (terreni e fabbricati, L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere i costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato italiano paralimpico per la partecipazione alla diciassettesima edizione dei Giochi paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per la celebrazione del Giubileo; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinarie già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 4-*bis*, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinarie svolte dal personale militare. L'articolo 5, comma 1, incrementa per il 2024 di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo, relativo al personale dell'area 5 della dirigenza per per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizioni di parte variabile dei dirigenti scolastici. L'articolo 6, commi 1 e 2, prevede delle disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie: si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu - Italia.

unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - A.U.S.A., l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati della finanza pubblica. L'articolo 6-*quater*, introdotto in sede referente, autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse i pagamenti degli interventi PNRR (comma 3). La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione L'articolo 6-*sexies*, introdotto in sede referente, prevede che i Ministeri, i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture vigente - e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Calandrini. Farò una sintesi della relazione, di cui depositeremo il testo per chi vorrà approfondire. reca disposizioni fiscali. L'articolo 7, al comma 1, come modificato in sede referente, consente anche ai soggetti che negli anni dal 2018 al 2022 dal 2018 al 2022 non abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA - stiamo quindi parlando del concordato preventivo biennale - a causa della diffusione della pandemia Covid-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote Irpef. L'articolo 7-*bis* consente a talune condizioni ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa. Il comma 1 dell'articolo 7-*ter* modifica la disciplina di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024: 2024: sopprimendo la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge, introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità. L'articolo 7-*quater*, introdotto in sede referente, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. L'articolo 7-*quinquies* limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale e della causa di cessazione del concordato relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, nei soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio associato. L'articolo 8 modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. 3, anch'esso introdotto in sede referente, dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda larga nelle aree bianche delle Regioni Lazio, Sicilia e Calabria. L'articolo 9 riconosce alla Regione Siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro nell'anno

in sede referente, stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670. L'articolo 9-*ter*, sempre introdotto in sede referente, abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione entro il termine prescritto dalla procedura di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali. L'articolo 9-*quater* modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e concerne i criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome del versamento da parte delle aziende farmaceutiche delle quote di ripiano a loro a carico (cosiddetto *payback*).

rappresentanti del Governo, colleghi, si continua a tergiversare sulle emergenze del Paese e, a questo punto, si rischia anche il baratro.

un'accozzaglia di misure eterogenee che non risolve i problemi economici e fiscali dei cittadini e delle imprese nonché degli enti territoriali. Si interviene sul rifinanziamento dell'indennità dell'Ape sociale - così come abbiamo ascoltato - ma si dimentica di renderla strutturale. La si finanzia solo fino al 2028, con risorse insufficienti: solo 27 milioni in media ad anno. La cosa più grave è che non si eliminano le discriminazioni nei confronti dei lavoratori che svolgono attività usuranti e che hanno una diversa aspettativa di vita. A questi lavoratori noi avevamo anche proposto delle correzioni, per riconoscere loro un'agevolazione di accesso all'indennità. Altro tema del provvedimento sono i Giochi del Mediterraneo. Qui il Governo e le forze di centrodestra si sono limitati a confermare i finanziamenti programmati dal Governo Conte II solo per le strutture sportive: 260 milioni. Ma il Governo e le forze di maggioranza hanno dimenticato i finanziamenti sulla mobilità e sui trasporti, oltre a quelli sulla rigenerazione urbana e sulla riconversione economica, sociale e culturale del territorio, dimostrando così completo disinteresse ai problemi e al rilancio della città di Taranto, ancora alle prese con il ricatto lavoro e salute. *(Applausi)*. I Giochi del Mediterraneo, pertanto, rischiano di ridursi a una semplice manifestazione sportiva di pochi giorni, senza cambiare il futuro del territorio. E si rischia anche che la manifestazione sportiva si svolga nel deserto, per l'assenza di collegamenti ferroviari, stradali e aerei. Altro tema in discussione è il lavoro straordinario già svolto dal personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Non si prevedono nuove risorse per gli aumenti salariali, per il rinnovo dei contratti e per la sicurezza. Preferite sprecare risorse per la missione in Albania, questa è la verità. Così come contro la criminalità dei colletti bianchi preferite cancellare l'abuso di ufficio. Inserite, poi, nel provvedimento in esame l'ennesima modifica del PNRR. Avete festeggiato, proprio qualche giorno fa, l'arrivo delle risorse. Siete abituati a festeggiare l'arrivo delle risorse, mentre nascondete la vostra incapacità nello spendere quelle risorse. *(Applausi)*. Siamo arrivati a meno di due anni

Solo nel 2024 avevamo 44 miliardi a disposizione, in base al programma che il Governo si era dato, e ne abbiamo spesi solo 9 su 44 per il 2028. alto è il rischio di restituire queste risorse, dimostrando così tutta la vostra incapacità. Eppure, eravate pronti a governare il Paese.

in esilio del ministro Fitto a Bruxelles. Infine, abbiamo altri temi. Innanzitutto, il bonus Babbo Natale: 100 euro per risolvere il problema della perdita di potere di acquisto dei salari del 15 per cento. Ma stiamo scherzando? Altro che bonus Babbo Natale: i lavoratori e i pensionati troveranno solo il carbone della Befana. Poi abbiamo la ZES Mezzogiorno, che è un vero disastro. Avete promesso alle imprese il 50 per cento del credito d'imposta. Lasciando le risorse invariate, quelle che erano state programmate, il credito di imposta che le imprese si sono trovate, anche in questo caso sotto l'albero di Natale, è appena del 18 State prendendo in giro tutta la classe imprenditoriale, nel silenzio più assoluto: questa è la vostra responsabilità. Adesso, pertanto, intervenite con un provvedimento vuoto di risorse. Vi è poi il concordato preventivo biennale: una misura annunciata come innovativa, uno strumento che doveva rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente contribuente e doveva basarsi anche sul contraddittorio; uno strumento che doveva garantire circa tre miliardi di euro da destinare alla riduzione della pressione fiscale sul ceto medio. nulla di tutto questo: è il fallimento annunciato di una misura vecchia di oltre vent'anni e spacciata per nuova. Questa è la dimostrazione che non avete un'idea innovativa. Come si fa a contrastare con questi strumenti vecchi di oltre vent'anni una evasione fiscale che supera gli 80 miliardi di euro l'anno? Con il fallimento di questo strumento cade anche l'obiettivo di ridurre le tasse al ceto medio, obiettivo che diventa così irraggiungibile. Anzi, l'Ufficio parlamentare di bilancio attesta che per il 2025 proprio quel ceto medio che è stato tartassato in questi anni rischia di avere una pressione fiscale in aumento, superiore al 50 Eppure, avete promesso di tutto per rimediare a questo fallimento annunciato: avete rinunciato alla progressività dell'imposta; avete introdotto un'imposta piatta del 10 e del 15 per cento, persino inferiore a quella proposta vent'anni fa dal Governo Berlusconi, che era del 23 e 33 È vero, pertanto, il detto per cui l'allievo ha superato il maestro, ma in questo caso vi siete veramente superati: avete esteso la misura anche ai contribuenti affidabili, minacciando persino i controlli. lasciamo in pace chi vuol fare! Questa è una misura coercitiva. Avete persino introdotto un condono fiscale per gli anni 2018-2022: il ventesimo in meno di tre anni. avete persino riaperto i termini, nella speranza di aumentare il gettito fiscale. Manca solo di offrire una vacanza *gratis* in un paradiso esotico, questo è ciò che manca! Pertanto, la riforma fiscale del Governo Meloni ha disatteso tutti gli obiettivi iniziali: non ha ridotto le tasse ai contribuenti, soprattutto al ceto medio; ha reso ancora più iniquo il sistema fiscale, creando diseguaglianze tra lavoratori e pensionati, da una parte, e e lavoratori autonomi, dall'altra; non ha semplificato la vita dei contribuenti; non ha contrastato l'evasione fiscale; non ha perseguito la redistribuzione della ricchezza; non ha tassato le nuove forme di ricchezza. In conclusione, il provvedimento in discussione rimane vuoto di soluzioni e non risolve nessuno dei problemi e delle emergenze: il PIL con una crescita dello zero virgola; la domanda interna stagnante; l'*export* che ancora perde non solo valori, ma anche volumi; una produzione industriale in calo venti mesi; precarietà; salari poveri; lavoro nero; evasione fiscale e contributiva; inflazione cumulata nel triennio del 17,3 A dimostrazione di tutto ciò, in conclusione, domani in oltre 40 piazze sciopera l'Italia che rivendica un diverso modello economico e sociale, a partire da un fisco equo, progressivo e proporzionale, con una reale capacità di redistribuzione della ricchezza, così come recita la Costituzione. Con questo provvedimento, quindi, il Governo Meloni

l'ho detto tante volte, ho una certa età, siamo senatori e mi sono stancato di ripeterlo, ma lo devo dire) - è l'ennesimo decreto-legge privo di elementi di urgenza e che si configura come decreto *omnibus,* nonostante i richiami del Capo dello Stato. Evidentemente questo Governo, visto che al secondo anno e quasi alla terza legge di bilancio del Governo Meloni, governa così. Non è una caratteristica dei nuovi arrivati, né una necessità dei primi mesi per prendere le misure, ma è un metodo, l'unico metodo che questo Governo conosce. Ed è un metodo nefasto. Non ha programmazione, non si confronta con la società e presenta documenti di grandissima frammentazione. Alla fine, siamo ormai alla produzione di decreti a mezzo di decreti. Come è stato detto

si sta cercando di capire dove possono essere queste persone. È un po' come in quelle aste e vendite dei mercati in cui, per convincere l'utente finale, si continua ad offrirgli qualcosa. Ormai è inutile chiamare ciò concordato preventivo. Cosa dovrebbe pervenire? Questo è un condono preventivo e un concordato successivo al fallimento del Governo. Qual è il guaio? A questa misura sono associati circa 2 miliardi di che, evidentemente, è inutile mettere all'attivo delle nostre politiche. Quindi, c'è non soltanto un fallimento del Governo, ma anche un serio problema di buco. Quando parliamo di buchi finanziari di questa entità, dobbiamo ricordarci che siamo in un quadro pluriennale, del Piano strutturale di bilancio, in forza del quale, se manchiamo un anno di equilibrio, dobbiamo ritrovarlo negli anni successivi perché va rispettata

L'insieme di queste misure, in particolare quelle del cosiddetto concordato preventivo, alla fine, diventando invece un condono preventivo, avranno un effetto fortemente dissuasivo, che già osserviamo, sulla fedeltà e fedeltà e *compliance* fiscale. Infatti se, alla fine, la rateizzazione o il ravvedimento operoso si realizzeranno comunque nel futuro, tutti quanti noi preferiremo posticipare

come quelle relative ai Giochi del Mediterraneo, al Comitato italiano paralimpico, al Giubileo e così via. Si tratta però di piccole spese che potevano tranquillamente non essere oggetto di un decreto d'urgenza, visto che stiamo approvando una legge di bilancio.

un'azione di verità: iniziamo a dircelo, iniziamo a raccordarci, questo Governo si raccordi con la Commissione europea per un'iniziativa che chieda la proroga delle scadenze PNRR. Questo Governo non riuscirà infatti a mantenere questi impegni. Ad oggi, su oltre 120 miliardi di spesa che dobbiamo realizzare, ne abbiamo occupati soltanto 30. Se guardiamo tutte le misure, gran parte di questi fondi devono essere spesi adesso con una strozzatura che evidentemente farà sì che noi non riusciremo a spenderli, li dovremo restituire, ma soprattutto metteremo una grandissima ipoteca sull'idea che le misure finanziate da debito comune europeo possano essere reiterate in futuro. Noi dimostreremo infatti di non essere in grado di rispettare quella spesa. Iniziamo adesso a prendere atto di questo elemento di verità. Iniziamo a chiedere una proroga alla Commissione europea; quello sì che è un provvedimento che si può fare. Tutto ciò che ha fatto il Governo sotto il profilo del PNRR fino adesso è stato semplicemente ritardare

altre questioni: torna la ZES unica. esattamente lì dove conviene che vadano, a meno di specifici incentivi. Se diamo incentivi a tutti allo stesso modo in un territorio, la parte che ne ha più bisogno non ne

ma sono ancora il 50 per cento di quelle necessarie. Ci sono molte lamentele dal punto di vista della soglia minima di accesso da parte di piccole imprese e artigiani, ma soprattutto, mentre si fa questo con la ZES unica, dall'altra parte, nella legge di bilancio si taglia il Fondo di agevolazione fiscale che fin qui è stato un elemento di grande impulso dell'economia del Mezzogiorno. Ieri Svimez ci ha detto che alla fine il saldo negativo per il Sud sarà pari a meno 5,9 miliardi. Avevamo delle misure complessive per circa 14 miliardi, avremo circa 6 miliardi in meno solo nel 2025 per il Sud. Da questo punto di vista, l'iniziativa di imposta sulla ZES non merita altri commenti. Si trovano inoltre risorse da togliere nell'assegno di inclusione; meno 200 milioni sull'assegno di inclusione. Ma come? Siamo qui a dire che c'è necessità di ridurre la povertà e le diseguaglianze, di sostenere le famiglie che hanno avuto più problemi per la spinta inflattiva, e togliamo risorse importanti a quell'assegno di inclusione del quale questo Governo si è molto vantato, ma che alla fine non è riuscito a coinvolgere tutti i soggetti necessari. E, poi, ancora, tagliamo dei fondi che servono a contribuire al bilancio della Commissione europea. Non mi sembra il modo migliore di avvicinarsi alle alle questioni europee in particolare. Infine introduciamo, tra le diverse modifiche, questo famoso *bonus* Natale, una misura già inaccettabile prima. Adesso lo si estende alle coppie di fatto, ma sostanzialmente questo importo non è minimamente capiente a coprire l'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie con redditi fino a 28.000 euro ed esclude completamente famiglie monoreddito, con redditi fino a 35.000 euro. Allora, quando si fanno queste misure (*bonus* Natale, *bonus* Befana e così via)

creare fondi di discriminazione. Per quanto riguarda il concordato preventivo, stupisce che si destinino 343 milioni di euro per coprire il debito della Regione Veneto per l'autostrada Il punto è che non soltanto sono risorse significative, ma questa copertura avviene con risorse tratte dal patrimonio destinato. Su questa vicenda abbiamo presentato un'interrogazione lo scorso anno, perché quella del patrimonio destinato fu una misura eccezionale, prima del PNRR, che adottò il Governo di allora per fronteggiare l'emergenza Covid. anno abbiamo chiesto in Commissione bilancio di avere informazioni sulla capienza residua di quell'operazione di patrimonio destinato, e ci è stato detto che su quel capitolo la cifra complessiva era zero e che si sarebbe esaurita con l'operazione che ha riguardato KKR e Telecom Italia. [**Presidenza

dei rappresentanti dell'opposizione, che per ben due volte hanno fatto passare la propria volontà bocciando proposte di legge di alcuni pezzi della maggioranza. Naturalmente in Aula è andato poi in onda

quel tipo di contrasto, vero o apparente, che abbiamo registrato non era su grandi questioni, non era sulla visione del futuro del Paese, non era sul rispetto o meno di una tensione programmatica, ma semplicemente su accordi accordi crepuscolari relativi ad interessi particolari. Quando avviene questo, vuol dire che c'è una crisi politica profonda perché il Governo del Paese non è basato su una forza coesa e su una visione comune di fondo, ma su accordi accordi che si succedono e che evidentemente in questo momento stanno scricchiolando. *(Applausi)*. Signora Presidente, colleghi, relatori, rappresentanti del Governo, quando fu ipotizzata la riforma della legge di bilancio che scorporava la parte fiscale dalla parte più generale, tale scorporo era volto a rendere palese e fare una fotografia reale della parte finanziaria, che rischiava, con l'antica legge di bilancio, di essere un po' annacquata nelle altre norme. Fu una riforma fatta dall'allora presidente Boccia, Governi Renzi e Gentiloni, che aveva questa finalità. Nel leggere questo decreto-legge fiscale a me manca la finalità, nel senso che l'avete fatto diventare un decreto *omnibus* dove sono previste regole e misure che non interessano il Paese o che comunque sono marginali.

all'interno di questa maggioranza. Non voglio essere spocchiosa: sia il centrodestra che il centrosinistra sono coalizioni che prevedono al loro interno delle diversità, e quindi, com'è toccato a noi dover mediare, toccherà giustamente a un partito di maggioranza come quello della presidente Meloni dover mediare con gli altri alleati. Voi forse siete più bravi a farlo nelle Aule specifiche e a non farlo sui giornali, come avviene invece per il centrosinistra; ma che questa maggioranza non sia unita lo si evince da tanti elementi. Innanzitutto un elemento di folclore che ha preso piede in tutti i decreti. All'inizio della legislatura c'era un solo relatore di maggioranza, adesso sono tre,

faccio notare quello che è successo ieri. A me fa piacere che Forza Italia abbia deciso di destinare le risorse che venivano tolte dal canone RAI

la sanità e la scuola, ad esempio, ma questo è chiedere troppo a Forza Italia. Però almeno ha dato un segnale del fatto che con le risorse pubbliche non si può scherzare. È vero che era uno sconto di 20 euro su una bolletta, ma

necessità; ricordo parole diverse quando c'eravamo noi al Governo, ma va bene ricredersi. Solo che le risorse sono poche. Continuare a rappresentare un Paese che sta bene, dove tutto va bene e dove le diversità sociali (la forbice) sono in continuo aumento è una cosa che non va bene, in primo luogo per voi che su questa narrazione avete vinto la campagna elettorale. Vorrei ricordare che, quando noi con orgoglio

voi ci rispondevate che quella era la finanza, erano brutali numeri, mentre il Paese reale faceva la fila alla Caritas. Ecco, ve lo comunico: il Paese reale continua a fare la fila alla Caritas. E con queste risorse,

l'inflazione ed è aumentato il costo della vita. Le famiglie normali, cioè quelle che hanno due stipendi in famiglia e che sono fortunate (forse non normali, ma fortunate, in questo periodo), non arrivano alla terza settimana del mese. Queste voi le avete dimenticate probabilmente negli *spot* emozionali che facevate durante la campagna elettorale; attualmente per voi non sono reali. aspetto che verrà ricordato, e non solo dai giornali di sinistra. Anche qui, dividere i giornali tra sinistra e destra lo trovo veramente incredibile, anche perché tutti hanno governato e tutti hanno ricevuto critiche. Allora non capisco: i giornali sono di sinistra o di destra a seconda di chi governa?

profonda divisione che arriva dalle ultime elezioni europee, che è continuata con le elezioni regionali e che andrà avanti, visto che le scadenze elettorali del prossimo anno sono ancora più numerose e riguardano Regioni a voi care. Tutte le Regioni sono a voi care, ma, se cito il Veneto, per un partito del Nord come era la Lega lo diventa molto di più (oppure la Lombardia). Insomma, ci saranno delle Regioni che voi volete tenere e confermare e quindi lo scontro all'O.K. Corral continuerà. Allora, ve lo chiedo perché ovviamente penso che gli spot elettorali emozionali, dopo due anni

parte delle opposizioni, che non per questo sono partigiane. Tutti noi riceviamo *e-mail* e sollecitazioni da portatori di interessi e di categorie sociali che chiedono maggior ascolto. Sono quelli che vi hanno votato, perché altrimenti non sareste qui a governare; non sono di sinistra o di centrosinistra, ma persone che dopo due anni di favole e di racconti di un mondo salvifico e meraviglioso, dove tutto funziona e tutto è roseo, incominciano a non poterne più, ma non ne possono più perché fanno i conti con la realtà, fanno i conti con i loro associati, che chiedono maggiore attenzione, fanno i conti con le liste d'attesa nella sanità, che continuano a essere enormi, fanno i conti con le emergenze. emergenze ambientali, i fondi sull'ambiente e sulla rigenerazione urbana sono inesistenti nella legge di bilancio che si sta discutendo alla Camera, come se queste alluvioni fossero un caso del destino cinico e baro e non fossero invece determinate da un cambiamento climatico che necessita di misure diverse e soprattutto di una diversa prevenzione, perché piangere sui danni e sulle vittime diventa veramente un esercizio di stile a cui le persone non hanno più voglia di assistere.

quando una società partecipa e vince un bando, avrà avuto i controlli del caso. Ora, mi dovete spiegare il senso della norma che prevede che nel collegio sindacale dei revisori dei conti, e delle finanze. Vi do questa notizia: neanche in Cina, nella Cina comunista, questo succede. E mi fa strano che chi ha parlato della bontà delle imprese e della capacità di fare impresa in questo Paese lo preveda. Allora delle due l'una: o a forza di andare da Musk e e in Cina siete diventati totalitaristi, oppure ricredetevi, perché vi do una notizia: quella norma è anticostituzionale.

nella Commissione bilancio su questo decreto. È ormai dall'inizio della legislatura che ne faccio parte e devo dire che

a licenziare questo provvedimento, non per volontà ostruzionistica delle opposizioni; anzi, abbiamo passato delle ore e delle giornate in cui non abbiamo discusso di nulla dal punto di vista del merito, ma abbiamo dovuto attendere

con cui cercavano di sbrogliare - non lo dico io, ma tutti i giornali ne hanno parlato in questi giorni - alcune contrapposizioni che stavano dentro

le parole della Presidente del Consiglio che, sul pasticcio della RAI, ha dichiarato che il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e di serietà. Ebbene, volevo capire quale decreto lei abbia letto

noi intervenissimo, ad esempio, rispetto al fatto che i salari continuano a perdere potere d'acquisto perché l'inflazione li erode, i contratti non vengono rinnovati, non c'è nessun meccanismo di recupero dell'inflazione e quindi, in sostanza, aumentano le disuguaglianze. Discutiamo,

c'è chi ha aumentato le proprie ricchezze, ma non viene toccato, anzi c'è un piccolo particolare: chi ha guadagnato molto non si tocca, all'incremento delle entrate dello Stato di circa 10 miliardi attraverso l'Irpef e grazie al fatto che lavoratori e pensionati continuano a pagare fino all'ultimo centesimo (e un giorno si stancheranno anche loro di farlo) voi introducete un concordato fiscale che non ha buttato quasi niente rispetto a quello che voi avevate previsto, perché avete dovuto ritirare la questione del concordato fiscale sperando di arrivare alla cifra che avevate ipotizzato, i famosi 3 miliardi circa, ma siete a

introducendo non la quinta rottamazione, ma andando oltre. In sostanza, è il contrario di quello che bisognerebbe fare,

alle manifestazioni e alle iniziative che si terranno nel Paese. Quelle iniziative, più che criminalizzarle, bisognerebbe ascoltarle, perché denunciano una sanità che non funziona

di sollecitare il Ministro, se c'è una risposta positiva o no. Sulla politica industriale siamo in una situazione in cui le crisi aziendali aumentano e non si vede la luce, perché, oltre alla Stellantis, c'è la Beko, c'è il petrolchimico, c'è tutta la vicenda di Siracusa, ci sono una serie di piccole e medie aziende. Quindi, è necessario affrontare questo

Signora Presidente, senatrici e senatori, questo decreto-legge, riguardante interventi di natura economica e fiscale, sta passando agli onori della cronaca come il campo di battaglia di uno scontro tutto interno alla maggioranza. I lavori della Commissione bilancio hanno registrato bocciature sonore e laceranti divisioni, che hanno dovuto far riflettere anche il Governo,

Non basta però buttare la polvere sotto il tappeto, perché questa situazione sta emergendo agli occhi delle italiane e degli italiani. In questo scontro tra i partiti della maggioranza abbiamo assistito a una guerra di tutti contro tutti.

Mi consenta, signora Presidente, una veloce precisazione su un elemento che ha sorpreso davvero tutti, cioè la questione del canone RAI. La prima osservazione: qualcuno spieghi che il canone RAI non è una tassa, ma il contributo dei cittadini e delle cittadine che posseggono televisioni e guardano i programmi della nostra RAI, affinché questo si realizzi. Continuare a parlare del canone RAI dicendo di tagliare le tasse è una bugia, signora L'anno scorso il taglio dei famosi 20 euro è costato 480 milioni alle tasche degli italiani e delle italiane, perché questa cifra è stata tolta dall'Erario, con le tasse pagate dagli italiani e dalle italiane (quelli che le tasse le pagano), e portata ovviamente verso la RAI, altrimenti quelle risorse mancavano ed erano indispensabili.

dai fondi di investimento di Ferrovie dello Stato: in un Paese dove ancora oggi abbiamo centri urbani caratterizzati dalla monorotaia, per finanziare l'emendamento che la Lega voleva, avremmo dovuto toglierli dagli investimenti della rete ferroviaria. Capisco che qualcuno se la canta e se la suona da solo, per cui da una parte si chiede di tagliare il canone

fosse invece emerso un voto favorevole all'emendamento presentato dal PD per ripristinare opzione donna, che ormai è stata talmente taglieggiata che l'anno scorso pochissime donne ne hanno potuto La passione per il taglio del canone, avrei voluto vederla lì, in un provvedimento che finalmente andava a favore delle donne lavoratrici del nostro Paese. Vi il tema del fisco, equo oppure non equo, direi il fisco iniquo; chissà che effetto farà

condoni e rottamazioni (uno, *bis,* *ter,* *quater*) ne sommeremo degli altri; loro non possono rateizzare; a loro nessuno chiede se ce la fanno a novembre o a dicembre a pagare le tasse. Si vedono poi le partite IVA poter rinviare, ancora una volta, sino a 170.000 euro. Non parliamo del giovane o della giovane partita IVA; parliamo

fisco equo, che manca drammaticamente nel nostro Paese? Tutta questa serie di rottamazioni e contraddizioni dentro al Governo diventa un invito all'evasione all'evasione e all'elusione fiscale. Altro che combattere l'evasione e l'elusione! E meno male che almeno vi siete fermati nel fare fare altre agevolazioni sull'evasione contributiva. Sarebbe stato troppo anche per voi, signora Presidente. Dobbiamo cambiare questo fisco per renderlo equo e avere un Paese dove vengono premiati gli onesti e non gli evasori e le elusioni. Per questo, signora Presidente, credo sia davvero ora di smetterla di prendere in giro gli italiani e le italiane. Avete fatto tante promesse, ma non ne state mantenendo una; anzi, state peggiorando le condizioni. Ho visto

DAL GOVERNO La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: - all'articolo 1, comma 6-*sexies*, le parole: "Anche al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies*" siano sostituite dalle seguenti: "al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies* e per le finalità di cui al terzo periodo";

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1274, di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo delle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. apre una nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155, nel testo proposto dalla 5a Commissione permanente, con le modifiche richieste

Signora Presidente, nell'iniziare questo mio intervento vorrei invitarvi a segnare questa data, il 28 novembre. Segnatevela, non tanto per i contenuti mirabolanti di questo decreto, in cui c'è poco e niente, ma perché io credo che con questa data inizierete a ballare la *rumba*. Questa maggioranza ha dimostrato che in questi giorni c'è stato l'avvio delle danze, delle difficoltà, delle incomprensioni

alcun risultato soddisfacente agli occhi degli italiani. Io me la segnerei la data ed eviterei di sottovalutare quello che è avvenuto in questi giorni in Commissione, quello che è avvenuto in questi giorni in Commissione, perché è avvenuto dopo alcuni passaggi politici molto importanti nel Paese: questa maggioranza ha perso le elezioni in due Regioni importanti, l'Umbria e l'Emilia-Romagna; vince le elezioni solo in Liguria, perché in Liguria il centrosinistra è andato diviso (lasciamo stare le responsabilità, non è questa e perché in quella Regione il contributo dei moderati e dei riformisti non è stato valorizzato. Il punto è che in Emilia-Romagna e in Umbria ci sono state sconfitte cocenti. Nessuno vuol far valere la dimensione di un voto regionale a questione di carattere nazionale, però secondo me c'è un campanello d'allarme e dobbiamo interrogarci sulle cause. Sono giorni molto complicati: pensate alla crisi dell'industria per quanto riguarda l'auto; pensate alla crisi dell'industria per quanto riguarda la moda; pensate al fatto che in questo Paese è una delle primissime volte che arriva un grido di dolore in piazza da parte di medici, infermieri e personale sanitario, non scioperano volentieri, perché in quelle professioni c'è un'etica, una visione di altruismo e di utilità e di utilità sociale che li porta a scioperare molto malvolentieri. Eppure in piazza ci sono andati per dire che la manovra di bilancio che sta per arrivare non affronta nessuna delle questioni centrali che riguardano la vita dei cittadini e una professione, come quella sanitaria, indispensabile alla vita dei cittadini. Allora quelle sconfitte, se le collochi dentro il contesto di difficoltà sociale che stiamo vivendo, con l'incapacità di questo Governo di aggredire il tema delle riforme in modo strutturale e serio e di provare a liberare risorse per le categorie, dal ceto medio a chi è fragile e debole nel nostro Paese, cominciano ad assumere, assieme a quei voti regionali, una dimensione di cambiamento di fase. Ora voi mi direte che non è così e che la Meloni è sempre popolare e che la Presidente del Consiglio continua a godere di consenso, ma quando arrivano sconfitte politiche, come quelle che ci sono state in Umbria e in Emilia-Romagna, significa che, pur mantenendo un livello di consenso, i problemi interni ed esterni a questa maggioranza cominciano ad essere particolarmente seri magari sono dati anche dal fatto che siamo passati dall'essere un Governo con una Presidente del Consiglio che era all'opposizione della maggioranza europea - di fatto - contribuire a quella maggioranza. Chi vi parla non ha avuto la postura, insieme alla forza politica che rappresento, di addirittura contro la Commissione e la vice presidenza di Fitto; al contrario, noi abbiamo sempre detto che tifiamo per il Paese e lo faremo fino in fondo, con il giusto e rigoroso atteggiamento istituzionale. significa che non ci è dato rilevare che voi avete fatto il gioco delle tre carte a scapito della coerenza con la vostra maggioranza e che oggi vi ritrovate in sede europea esattamente all'opposto di come avete dichiarato ai cittadini durante le elezioni europee. Questi sono temi che prima o poi vengono a galla.

Poi infarcite questo decreto nel corso dei lavori di una serie di questioni che riguardavano gli enti locali. Provate a convincere la minoranza - che con atteggiamento istituzionale collabora, cerca di dare una mano, sente l'ANCI, si fa carico di alcune istanze importanti anche nel mondo degli enti locali - che quella sarà la vera partita nella quale provare a dare segnali di accettazione di alcuni temi giusti. Poi però, in corso d'opera, fate carta su, non rimane niente di quel decreto e tagliate tutti gli emendamenti che l'opposizione ha portato, ma nonostante ciò non riuscite a uscire dalle difficoltà. Non ce la fate perché arriva un emendamento da parte della Lega sul tema del canone RAI. Su quell'emendamento si articolano i pizzini di cui parlavo prima, per varie ragioni, all'interno della maggioranza e andate sotto andate sotto in una polemica palese, pubblica, che significa che a voi, anche del tema della RAI

ma arrivare senza una proposta di riforma, solo ed esclusivamente per regolare i rapporti e i conti interni alla maggioranza credo che sia stato davvero - lasciatemelo dire - demenziale. Ma non è finita lì, perché, a seguito del fatto che Lega e Forza Italia si sono praticamente accapigliati sul tema della RAI, è arrivata la vendetta, che ha colpito - ahimè - Occhiuto, Occhiuto, che aveva bisogno di avere un emendamento di Forza Italia sul tema della sanità e dello sbilancio nella sua Regione un po' complicata dal punto di vista sanitario (e non solo nell'ultima fase di Occhiuto, ma per tradizione), e che si vede bocciare dalla sua stessa maggioranza un emendamento che aveva costruito con Forza Italia. La cronaca la conoscete, perché i giornali li leggiamo tutti, ma io vi voglio sottolineare perché è avvenuto ciò. È avvenuto non solo perché siamo in presenza di un decreto che non dice nulla, che non aiuta una categoria italiana, che non è una proposta di revisione del fisco, ma banalmente un'accozzaglia di elementi senz'anima e senza visione; perché quella capacità di cucitura, quella funzione di cerniera, quella capacità di governo della maggioranza che era propria di Fratelli d'Italia comincia a scricchiolare e scricchiola non solo perché premono Salvini e Tajani, ma banalmente perché i conti in tasca agli italiani cominciano a non tornare: non tornano quando si promette loro di aumentare le pensioni minime e poi gli aumenti sono di 3 euro, non tornano quando sulla sanità non viene data una risposta e quindi medici e infermieri vanno in piazza a lanciare il loro grido di dolore, non tornano quando si fanno i decreti sulle liste d'attesa, ma questi non servono a niente.

al collega Lupi, nella quale viene posta una domanda: l'apericena costruito dalla Meloni per trovare una sintesi anche in vista della legge di bilancio, che sarà soltanto l'antipasto (a proposito di metafore culinarie),

sempre l'acuto Lupi in qualche modo mette in evidenza è che ci sono sempre state le divisioni nella sua maggioranza, ricordando quando il presidente Berlusconi metteva insieme Bossi

immediatamente prima della legge di bilancio, vi inviterei a considerare tale giorno come una data nella quale davvero inizierà la rumba. Vediamo dove ci porterà. Quello che io vi posso dire è che troverete questo fronte del campo, magari non allineato su tutte le proposte, ma

gravissima, cioè la situazione economica che abbiamo ereditato. Noi stiamo tentando in ogni modo di portare avanti dei provvedimenti molto pragmatici,

di là dei provvedimenti del cosiddetto decreto fiscale - elemento fondamentale di quella che sarà la manovra finanziaria, dove andremo a toccare argomenti come le risorse per l'efficientamento delle reti ferroviarie oltre 30 milioni per mettere in bella mostra quella che è l'Italia agli occhi del mondo per quanto riguarda gli eventi internazionali sui nostri territori, come le Olimpiadi e i Giochi del Mediterraneo a Taranto, importantissimi, in una città che ha sofferto e soffre ancora, da anni, una situazione particolarissima. Oppure, penso ai Giochi paraolimpici.

Mettiamo in campo delle risorse per far sì che il PNRR possa avere una immediatezza per quanto riguarda le capacità di erogazione dei fondi, soprattutto per chi dovrà realizzare i lavori, così da non far trovare in difficoltà le aziende

con maggiori difficoltà di carattere economico e di conseguenza sociale di comprare un giocattolo in più ai propri bambini. Quindi, si amplia la misura a tre milioni di persone, di famiglie che potranno usufruire di questo piccolo sostegno. sostegno. Il taglio dell'Irpef ci è consentito grazie al concordato preventivo biennale, alla proroga che c'è stata, in modo tale da poter intervenire soprattutto sul ceto medio. Se poi anche i giornalisti economici di "la Repubblica" imparassero a fare i conti e leggessero bene quali sono i prelievi da fare al ceto medio, magari sarebbe più facile spiegare ai cittadini che non si sta facendo una misura con l'inganno e che, se si abbassano le percentuali, diventa difficile

che, per poter uscire dalla situazione nella quale ci trovavamo dal punto di vista economico, ci vorrà ancora del tempo. Tuttavia, tutti i parametri economici vanno in un'unica direzione, quella della crescita

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare andrà a sostegno di una manovra che continuerà sulla linea che abbiamo intrapreso e, a differenza di quello che ci viene detto,

deve essere in grado di affrontare le differenze in modo politico e, quindi, confrontandosi. Invece vi nascondete, perché siete talmente divisi e continuate a litigare, che decidete

quali prebende vanno a Tizio o a Caio. Questo è ciò che fa scattare la tensione. Quindi, bisognerebbe prendere atto di questa difficoltà, magari non

La cosa insopportabile di questo decreto è il messaggio che viene dato agli italiani: se fai il furbo, hai la possibilità di continuare a farlo, anzi sarai premiato. Questo è il dato. Se fai il furbo e non paghi le tasse, sarai premiato.

Se volete vi porto una busta paga che ho e vi dimostro che la voce della scala mobile era più alta della paga base del contratto.

È un modo per affrontare la questione dei bassi salari il fatto che ci siano 4 milioni di persone che prendono meno di nove euro lordi l'ora? Quelle

non è quella la strada percorribile. Non è pensando di premiare chi non paga che noi risolviamo il problema. Anzi, facendo così, aumentiamo la voglia di non pagare. Per queste ragioni, in sostanza, bisogna invertire la tendenza. Noi assistiamo sostanzialmente al fatto che anche in questo decreto-legge, legato alla legge di bilancio - che è la legge più importante che dovrebbe affrontare i problemi

perché mette in campo impegni di spesa che dagli iniziali un miliardo e 740 milioni sono diventati due miliardi e 340 milioni. Il bilancio dello Stato è cresciuto a dismisura tra il 2019 e il 2022, anche a causa delle misure straordinarie richieste, prima per affrontare l'emergenza pandemica poi, la crisi economica conseguente, a cui si sono aggiunti gli interventi per aiutare imprese e famiglie a superare l'aumento del costo dell'energia a causa del conflitto russo-ucraino. Il bilancio dello Stato viene ricondotto ora a cifre più ragionevoli, ma soprattutto si torna a investire attraverso una puntuale operazione di riqualificazione della spesa. Il fatto più evidente di questo decreto-legge è la revisione della spesa corrente a carico dei Ministeri per un miliardo e 740 milioni di euro, andando a individuare sprechi e sovrapposizioni. Il Piano strutturale di bilancio, nel rispetto delle nuove regole europee, punta a una graduale, ma sostanziale diminuzione del ricorso della spesa in *deficit* sulla strada della sostenibilità dei conti pubblici. Ne consegue la necessità di una riqualificazione della spesa pubblica e di un maggiore sostegno agli investimenti per far ripartire l'economia a sostegno del PIL. Mettere in ordine i conti pubblici, spostare fondi dalla spesa improduttiva al sostegno della produzione, incentivare gli investimenti e, al contempo, sostenere il potere di acquisto delle famiglie sono gli obiettivi della manovra nel suo complesso, cui questo decreto dà il proprio contributo. Si parte dagli investimenti nella rete infrastrutturale delle Ferrovie dello Stato e dagli investimenti sulla rete stradale di competenza di ANAS, che assorbono il grosso degli impieghi del provvedimento. Il recente blocco delle stazioni ferroviarie di Roma Termini e di Roma Tiburtina riporta in evidenza la necessità di ulteriori investimenti sulla rete ferroviaria, diventata fondamentale di fronte a un numero di viaggiatori crescente che sceglie di viaggiare in treno. In questo senso vengono stanziati 750 milioni di euro a Rete ferroviaria italiana e 300 milioni alla infrastruttura ferroviaria. Allo stesso tempo, la rete stradale nazionale gestita da Anas, che si è arricchita di nuove tratte, ha evidenziato l'esigenza di ulteriori finanziamenti per essere mantenuta e ammodernata. Si tratta di ulteriori contributi all'infrastrutturazione, di cui 300 milioni destinati ad Anas e 343 milioni per rafforzare la dotazione patrimoniale di Autostrade dello Stato. Inoltre, il decreto contiene disposizioni per semplificare ulteriormente la realizzazione delle opere con il PNRR, prevedendo la riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni centrali e locali. Sempre in funzione di ulteriori investimenti sul territorio vengono inoltre riconfermate alcune misure, come il sostegno di 25 milioni di euro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto; milioni di euro per i Giochi paralimpici del 2024; a Roma Capitale che è diventata ormai da mesi un grande cantiere per affrontare il grande Giubileo del 2025, vengono assegnati ulteriori quattro milioni. Insomma, si mette in campo un sostegno ulteriore e concreto agli investimenti e all'infrastrutturazione, che anticipa, in quanto contenuta nel decreto-legge già vigente, quel piano di investimenti previsto anche dalla legge di bilancio 2025. Viene nuovamente e giustamente riconosciuta da parte di questo Governo l'importanza delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del personale militare, a cui va un contributo di 120 milioni per remunerare il lavoro straordinario che viene riconosciuto agli operativi. Il personale in divisa affronta sacrifici quotidiani di fronte alla necessità di ulteriori controlli del territorio e all'esigenza di percepire maggiore sicurezza che viene richiesta dai cittadini. La Commissione bilancio del Senato ha inoltre apportato una serie di modifiche, innanzitutto la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale. Il concordato-*bis* guarda agli indecisi che non hanno aderito alla prima *tranche*; si applicano le stesse condizioni e il termine ultimo è fissato al 12 dicembre. Viene anche ampliata la platea del *bonus* Natale da 100 euro. È stato inoltre stabilito il rinvio dell'acconto delle tasse per le partite IVA, che potrà essere pagato anche in cinque da gennaio a maggio 2025. È un decreto-legge su cui la maggioranza ha adottato le disposizioni necessarie per sostenere la crescita del Paese. Pensate che in soli due giorni questa maggioranza, tra Camera e Senato, ha approvato compattamente lo stop al numero chiuso a medicina, il decreto flussi e oggi il decreto fiscale. A fronte di tante novità, provvedimenti e investimenti per il nostro Paese, c'è chi si sofferma solo sulla questione dell'emendamento sul canone Rai. Noi riteniamo che ridurre agli italiani il canone di 50 centesimi al mese a testa non abbia un grosso impatto. Se poi si considera che lo Stato deve prendere 430 milioni dalla fiscalità generale per darli alla Rai al fine di sopperire al taglio del canone, si capisce che per noi sia una proposta meno efficace di altre. Forza Italia ritiene che sia prioritario continuare nella politica di riduzione delle tasse intrapresa dal centrodestra. A tal fine, rilevato che c'era la disponibilità di 430 milioni che sarebbero stati destinati alla Rai, proponiamo che questa cifra venga destinata a un fondo per tagliare l'Irpef, a tutela dei ceti medi in particolare. Aggiungendo a questi 430 milioni i proventi del concordato fiscale, che è stato opportunamente prorogato dalla maggioranza di Governo proprio in questo provvedimento, si potrà ottenere una cifra superiore al miliardo, che potrà contribuire a tagliare le aliquote Irpef. Abbiamo già confermato e stabilizzato il taglio del cuneo fiscale e a altri provvedimenti che aumentano il reddito netto delle famiglie. Con un fondo taglia Irpef daremo un ulteriore segnale concreto. Partiamo da questi 430 milioni e chiediamo al MEF di vincolarli a questo obiettivo, in attesa di avere a disposizione altre risorse. Tagliare le tasse è la priorità di sempre di Forza Italia. Rispetto a quanto è successo, vi voglio dire che noi rispettiamo le idee della Lega e sono sicuro che i colleghi leghisti rispettino le nostre. Così si vive in una grande famiglia come il centrodestra: non il pensiero unico, ma il confronto. La stragrande maggioranza delle volte il confronto porta a una veloce sintesi; poche altre volte ciò non accade e si discute un po' di più. Ma oggi siamo più forti e coesi, perché sappiamo che approviamo un provvedimento importante, l'ennesimo nella giusta direzione per rendere più forte il nostro Paese; una manovra di bilancio nel suo complesso, come ha certificato ieri anche la Commissione europea, che si muove in un ambito virtuoso di messa in ordine dei conti pubblici, generando indicatori di crescita apprezzabili. Sono segnali in linea con le previsioni del Governo, che erano prudenti e che potranno quindi essere superate da dati anche più favorevoli. Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia danno il loro convinto voto favorevole al decreto e alla fiducia. E chi vuole - Presidente, mi rivolgo ai colleghi per suo tramite - si crogioli pure nell'illusione di maggioranze che si sfaldano. Nel frattempo noi di centrodestra continuiamo a governare efficacemente il Paese negli interessi degli italiani.

ogni tanto vorrei essere a corto di argomenti per commentare o criticare le azioni del Governo e della maggioranza. Ma devo dire che - ahimè, ahivoi - mi date sempre fin troppo materiale e mi rendete il lavoro particolarmente facile, a volte persino divertente. Come in questo caso, dove abbiamo due decreti confluiti in uno che fanno una sola cosa, più che evidente: certificare la vostra totale incapacità in materia economica. Non sapete più da che parte e in che modo arrabattarvi per cercare di risolvere i problemi che avete creato voi stessi, come per esempio il famoso e così decantato concordato fiscale preventivo, che era talmente appetibile che hanno aderito così pochi che siete stati costretti a riaprire i termini. Non è che sia andato favolosamente e, quindi, l'avete riaperto ancora un po' per accontentare quelli che, indecisi, erano rimasti un attimo indietro e poi vi hanno suonato per dire: «Ohi, ohi, voglio partecipare anch'io a questa cosa bellissima!». non è andata così. È andata che non vi si è filati nessuno e, quindi, avete disperatamente riaperto i termini, con un allargamento del ravvedimento operoso, leggasi condono, che pure quello ormai non piace più nemmeno agli evasori; cioè nemmeno alla vostra platea di utenti favorita riuscite più a parlare, perché pure quelli vi snobbano. Avete tentato *in extremis* di riaprire i termini, cercando di convincere qualche milione di riottosi, perché sono tanti quelli che non hanno voluto aderire.

e lo certifica quello che c'è scritto in questo decreto. Quindi un altro fallimento, un'altra promessa tradita. E voi eravate quelli bravi, ma complimenti! Ogni tanto riuscite pure a rimediare a qualche errorino fatto per strada, come nel caso del *bonus* Babbo Natale. Avevamo detto in questa stessa Aula che era semplicemente un anticipo e che era pure fatto male, perché tagliavate fuori tantissimi potenziali beneficiari, che avevano i requisiti di reddito, a cui volevate elargire il bonus; ma avevate messo le maglie troppo strette e, quindi, quei soldi non sarebbero arrivati. Noi vi avevamo suggerito con numerosi emendamenti in quel provvedimento come risolvere il problema e praticate il vostro sport preferito: il furto dell'emendamento. Quindi, avete respinto come sempre tutte le proposte delle opposizioni e poi quello che avete cacciato dalla porta lo fate rientrare dalla finestra nei testi dei vostri emendamenti, a firma del Governo o dei relatori, quello che sia, tanto ormai non c'è più distinzione. Ebbene, Ebbene, accontentate - si fa per dire - qualcuno in più, cosa su cui ovviamente non abbiamo assolutamente nulla in contrario, però dovete dire che avete "spintaneamente" fatto quello che vi era stato chiesto da altri. da altri. Che cosa abbiamo visto in questo provvedimento, oltre all'evidente incapacità della maggioranza e di chi ci governa? Abbiamo visto che questo clima di compattezza granitica della maggioranza comincia a mostrare crepe tutt'altro che lievi: Forza Italia vota contro l'emendamento della Lega per la riduzione del canone Rai; la Lega si vendica con delle astensioni e non votando l'emendamento di Forza Italia sulla sanità calabrese, che voleva sanare *a posteriori* bilanci - diciamo così assistiamo alle ripicche, mentre aspettiamo ore e ore estenuanti in Commissione che qualcuno si decida a dirci di che morte deve morire questo Paese con siffatti incompetenti alla guida. Di sicuro c'è una cosa: la Lega sa benissimo chi sono i suoi interlocutori preferiti e preferenziali. Da una parte ci sono la Lombardia, il Veneto e le Regioni del Nord, quando si oppongono alla ripartizione del *payback* dei farmaci con la finta storia che sicuramente dopo di me l'illustre professore Garavaglia, economista, saprà spiegarvi meglio della povera biologa che non capisce niente di economia. Quello che ho capito è che la Lombardia con degli *escamotage* mette a carico di capitoli diversi di bilancio alcuni farmaci più costosi, perché le cure sono fatte da istituti privati e vengono rimborsate su capitoli diversi da quelli della spesa diretta dei farmaci che le altre Regioni, che si avvalgono prevalentemente della sanità pubblica, fanno su quei capitoli di bilancio su cui poi si calcola il *payback*, e però poi partecipa alla ripartizione dei soldi che arrivano indietro dalle imprese farmaceutiche. Quindi, vogliono fare i primi della classe con un *escamotage* e poi sono dispiaciuti quando le altre Regioni li beccano con le mani nella marmellata e cominciano a dire che magari le cose devono farle in maniera più equa. Poi, altro interlocutore preferenziale, soprattutto a leggere gli emendamenti firmati dal senatore Garavaglia, sono gli intermediari finanziari, a cui volevano regalare - a mio umile avviso - i cinque miliardi dei cittadini italiani che hanno dei contenziosi aperti per la restituzione delle spese accessorie, quando estinguono anticipatamente una cessione del quinto. E invece, stoppando l'emendamento, i contenziosi restano in essere e i soldi restano ai cittadini. Anche su questo il collega sicuramente ci illuminerà, ma io ve lo spiego, come la capirebbe la signora Pina che fa l'operatrice La signora Pina, cinque anni fa, ha fatto una cessione del quinto dello stipendio per pagare le spese dentistiche del figlio. Quando ha aperto il finanziamento della cessione, ha pagato in anticipo un'assicurazione sulla somma che le è stata erogata valevole per dieci anni e in alcuni casi ha pagato in anticipo pure le spese di riscossione della rata. Dopo cinque anni ha avuto - ahimè, per lei - un'eredità dai genitori e ha estinto anticipatamente la cessione. Ha diritto, in base alle leggi europee, a riavere indietro quello che ha pagato in anticipo per i cinque anni in cui non pagherà le rate e non usufruirà, quindi, dell'assicurazione; quei

Insomma, signor Presidente, mi sembra evidente che questa sia l'ennesima dimostrazione del vostro totale fallimento in materia economica di dire che avete ereditato una situazione difficile a causa dei buchi - non esistono - nel bilancio dello Stato creati da noi. Quando vi abbiamo lasciato le chiavi della macchina, la macchina stava viaggiando bene. Magari aveva bisogno di un'aggiustata a qualche bullone, ma sicuramente non perdeva pezzi. Quelli glieli avete fatti perdere voi, perché non siete rimandati a settembre, siete bocciati su tutta la linea, come bocciato dovrebbe essere questo provvedimento. *(Applausi)*.

Signora Presidente, preannunciando il voto favorevole della Lega a questo provvedimento, nel salutare le colleghe senatrici e i colleghi senatori, inviterei a cercare di fare qualche approfondimento su quanto abbiamo approvato. Il decreto fiscale - come sappiamo - è di fatto la base della legge di bilancio, la quale ha una caratteristica,

questa è per noi una faccenda di principale importanza. Inoltre, è una legge di bilancio coerente con le nuove, vecchie regole europee. regole europee. Con le nuove regole europee, siamo tornati alla normalità: per fare una spesa, bisogna trovare una copertura. Dopo anni di sforamenti miliardari in via eccezionale - prima c'erano le crisi finanziarie, poi c'è stato il Covid - adesso siamo alla normalità: fai una spesa, la copri. In più, la spesa è sotto controllo: nei prossimi cinque anni, mediamente, la spesa corrente non può crescere più dell'1,5 Tenendo conto dell'inflazione, sostanzialmente bisogna stare a zero *budget*. Tenendo conto del fatto che alcune voci di spesa crescono autonomamente - come le pensioni, per via della piramide demografica va da sé che vanno fatte delle scelte, ci saranno voci che crescono anche meno (di zero) e voci invece su cui si investe. In particolare, si investe sulla sanità - checché se ne dica - che è una delle poche voci che va a crescere e cresce più di quel famoso 1,5 Non è un caso che poi la manovra sia stata promossa dalle strutture europee, cosa che è stata direi poco pubblicizzata e poco nota. Rispetto ad altri Paesi che hanno che hanno avuto invece un tratto di penna rossa sulle loro leggi di bilancio, l'Italia ha avuto un parere positivo. Ma soprattutto è stata promossa dai mercati, che tengono sotto controllo i nostri tassi di interesse e hanno ridotto lo *spread*. Questo fattore dei tassi di interesse è fondamentale, perché in futuro vedremo anche una diminuzione della quota base del tasso dovuta alla riduzione del tasso che farà la Banca centrale europea, ancorché con un certo ritardo. Questa riduzione ci sarà e sarà importante. Però, è importante quello che dipende da noi, che è proprio lo *spread*. Quindi, la credibilità paga, ma anche la stabilità politica paga. Su questo la Lega è molto attenta ed è un pilastro solido di questa maggioranza proprio in termini di stabilità, perché la stabilità politica L'Italia non è più il malato d'Europa, ma bisogna proseguire con attenzione su questa strada. Non possiamo permetterci incidenti di percorso. Nel decreto fiscale, abbiamo

Inoltre, grazie alla Lega, è stata riproposta la rateizzazione dell'acconto. Sapete che l'Italia è un Paese strano. L'Italia fa pagare in anticipo alle partite IVA le tasse dell'anno dopo: il reddito lo produci l'anno dopo, ma paghi le tasse l'anno prima. È una cosa ovviamente demenziale, ma è così. abbiamo iniziato questo percorso che consente di spostare in parte il pagamento delle imposte nell'anno in cui si genera il reddito con cui pagare queste imposte. Lo abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo riproposto la misura quest'anno. L'idea della Lega è di renderla una misura strutturale e allargare ancora di più questa possibilità, affinché sia disponibile per tutte le aziende. C'è però un problema, relativo alle risorse. Tutti, infatti, parlano di una legge di bilancio di 30 miliardi, ma in realtà non è vero. La legge di bilancio è di 60 miliardi,

Tutto bene, ma, come sempre, ci sono dei problemi. I problemi, però, vanno risolti e non vanno fatti esplodere. Per noi della Lega, i problemi vanno risolti. La politica è mediazione e soluzione di problemi. È l'arte dell'impossibile.

Evidentemente ad un maggiore sforamento: questo è pacifico. Siccome il *payback* è una tassa sulle aziende che producono farmaci, va da sé che fare una norma che aumenterà lo sforamento negli anni prossimi porterà all'incremento di queste tasse alle aziende. Ne abbiamo già sentita qualcuna. Questo porterà, evidentemente, ad una riduzione degli investimenti, italiani ed esteri, in questo settore che è strategico per il nostro Paese. Ci auguriamo che ci sia un ripensamento. Sono certo che ci sarà e che si troverà una soluzione diversa, perché risolvere un problema creandone uno molto più grande non è una trovata geniale. Concludo con una considerazione sul concordato fiscale. Una delle critiche al concordato fiscale è che finora vi aderiscono le aziende che ne avranno un vantaggio e quindi pagheranno meno tasse. Bene, la Lega è per far pagare meno tasse. *(Applausi)*. Noi siamo convinti che, a parità di spesa, la spesa fatta dal settore privato produce più PIL della spesa fatta dal settore pubblico. Questa è una certezza matematica. È così. Quindi, noi noi siamo convinti che la credibilità e la stabilità di questo Governo siano il vantaggio competitivo del sistema Paese. I mercati lo stanno vedendo e ci stanno premiando.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, le difficoltà della maggioranza nella conversione del decreto-legge fiscale sono apparse evidenti, non solo ai mezzi di informazione, nelle giornate di ieri e di oggi. Per chi le ha vissute direttamente, mostrano una maggioranza allo sbando, senza nessun livello di tenuta, con priorità che non si connettono tra di loro. Se uniamo il disastro di ieri al voto della Lega nel Parlamento europeo, contrario alla Commissione che ha come Vice Presidente un Ministro della vostra maggioranza e della nostra Repubblica, direi che non solo l'Italia è priva di un piano strategico per il futuro del Paese, ma non avete alcuna idea nemmeno rispetto a come costruire un'Europa utile ad un nuovo progetto di sviluppo industriale. È evidente che tutto questo segna uno spartiacque anche in questa legislatura, perché non c'è dubbio che avete concluso il tempo utile della vostra luna di miele; si è consumata definitivamente, anche esternamente, la vostra immagine (che era più nella propaganda) di solidità, di infallibilità; l'idea, cioè, che avete una tenuta solida, che perfino non richiede la costruzione di un'alternativa di Governo. Questo è il motivo vero per il quale io credo che nella giornata di ieri si sia consumata una prima parte fallimentare della vostra legislatura. Oggi emerge con forza la necessità di costruire un'alternativa; c'è una responsabilità anche nostra - dopo ne dirò - relativa al fatto che stiamo cercando, di fronte ad ogni decreto-legge in conversione, di introdurre, attraverso emendamenti alle proposte legislative, la consapevolezza di un'idea di Paese che abbiamo in testa che è diversa dalla vostra. Tuttavia - lo dico al netto della vostra propaganda e di una vostra capacità di rappresentare in esterno la vostra autorevolezza - io penso che siate bloccati dall'insostenibile principio: una cosa a me, una cosa a te; cose che spesso, peraltro, sono in contrapposizione e che non vi consentono di trovare il filo di un'idea dello sviluppo del Paese, di come contrastare la povertà, la solitudine, del come garantire lavoro e crescita economica. Dico questo perché, se ci pensiamo bene, avete avviato il processo dell'autonomia differenziata, che con il premierato non c'entra nulla, anzi sono due follie istituzionali, insieme all'attacco insostenibile al pilastro della giustizia. Il fatto che nell'accordo di Governo abbiate una cosa per ciascuno rappresenta un danno per tutto il Paese, per i lavoratori, per le famiglie, per i giovani, perché non garantisce alcuna prospettiva. Queste sono le vostre riforme, che sono tutte su un binario morto e sono fortunatamente tutte bloccate nelle vostre divisioni e frammentazioni. Il decreto-legge fiscale non è un decreto-legge ordinario; è la base, come veniva ricordato dal collega Garavaglia, di una legge di bilancio, dunque siamo in presenza di un evento grave su un provvedimento importante, perché la maggioranza ha dimostrato anche di non avere i numeri per approvare, con il parere favorevole del Governo, le vostre contraddizioni irrisolte.

a botte di ravvedimenti, concordati, proroga termini; avete inquinato il pilastro del sistema fiscale, della progressività e della fedeltà attraverso processi di *flat tax* che di fatto caricano oneri fiscali crescenti (non calanti) sul lavoro dipendente, sulle pensioni. È l'esatto contrario di quello che serve sul versante della progressività e dell'equità sociale. State contribuendo a far passare un'idea, attraverso i fallimenti delle previsioni di bilancio, perché per voi il concordato è il fazzoletto sotto il quale nascondere le entrate che non ci sono.

e voi li state accompagnando, a proposito di equità e fedeltà fiscale, verso un privilegio che riguarda le fasce alte della fedeltà fiscale.

sono qualcosa di inutile (tanto arriverà, sempre di più e sempre prima, un Governo di destra che alla fine introdurrà un condono, un *escamotage*) e state anche creando un danno sulla progressività e sull'equità, che è un pilastro del sistema fiscale. Ieri avete toccato il massimo in tutto questo. Pensiamoci bene e con attenzione. Ieri siete addirittura riusciti nel capolavoro di confondere un canone con una tassa.

viene pagato in base a un servizio che mi viene erogato. Il canone Rai lo paghiamo perché c'è un servizio pubblico che arriva nelle nostre abitazioni. La tassa, anche se non uso i servizi, la pago ed è quindi cosa diversa dal canone. Avete pensato di abbassare di 20 euro il canone, con il consenso di Fratelli d'Italia e immagino anche della Presidente del Consiglio, utilizzando 430 milioni di RFI, di RFI, per nascondere che ci sono 430 milioni di oneri per la finanza pubblica a carico dei lavoratori e dei dipendenti. *(Applausi)*. Ancora oggi state sostenendo questa misura come utile,

perché sono follie. Abbiamo lavorato affinché questa cosa non accadesse, perché sarebbe stata dannosa per i lavoratori e i pensionati di questo Paese. Paese. Aggiungiamo poi la farsa del ministro Salvini, che ha fatto questo decreto dove, al comma 1, incrementa di 250 milioni di euro il RFI e aggiunge altri 750 milioni per finanziare il contratto di programma. Voi volevate comunicare la riduzione della pressione fiscale fermando treni che sono già in ritardo. Ma che idea di Paese avete? faccia il Ministro e stia sulle sue funzioni fondamentali, che sono quelle di garantire un trasporto pubblico efficace; non usi questi *escamotage* per caricarsi di responsabilità che non gli competono.

Non avete fatto alcun investimento sulla formazione, in termini di risorse umane, sulla scuola, sull'università e sulla ricerca. Non avete uno straccio di piano per lo sviluppo industriale ed economico dell'Italia. Abbiamo presentato due emendamenti per provare se la vostra propaganda resta nel programma di mandato. Il primo è quello su Opzione donna: l'avete respinto, respinto, negando l'opportunità di affermare una delle più grandi questioni di genere, interessanti e indispensabili, per favorire l'uscita delle donne dal sistema del lavoro in maniera più giusta. Avete detto di no alla proroga al 31 Siete riusciti a dire di no al contratto di apprendistato, l'unica forma che consente ai giovani di poter uscire ed entrare nel mondo del lavoro senza il ricatto dello *stage* gratuito. *(Applausi)*. Avete detto di no a questioni che servono all'Italia e avete detto di no a questioni che, per quello che ci riguarda, consentiranno a noi di lavorare nel Paese per preparare un'alternativa a questa destra che non è in grado oggi di corrispondere alla fiducia che questo Paese merita nei confronti di un Governo. Per questa ragione votiamo no alla fiducia.

Testor, Damiani e, in particolar modo, alla collega Ambrogio, che non vedo in Aula, per tramite anche del sottosegretario La Pietra, a tutto il Governo. Vedo Lucia Albano, che ha seguito i lavori, il ministro Giorgetti e saluto, in particolar modo,

prezioso provvedimento il nostro, come abbiamo detto in tanti in quest'Aula, perché è prodromico, complementare e anticipatore della legge di bilancio.

rapida ricordo i passaggi più importanti: il concordato biennale che è stato esteso in termini di data fino al 12 dicembre; il *bonus* Babbo Natale, che avete avete combattuto perché non abbastanza esteso come platea, è stato esteso da un milione di persone (questa era la platea di riferimento) a 4,5 milioni di genitori *(Applausi)*, quelli che voi auspicavate venissero coinvolti. attenzione sulle liste d'attesa, sulla protezione civile, sul rifinanziamento dell'APE sociale. Sono state previste misure per i tempi del PNRR con interventi sulla piattaforma Regis. Capisco che molti non sappiano neanche cosa sia una piattaforma Regis *(Applausi)*; questo è il problema che avete con i vostri rappresentanti territoriali. Lo dico guardando il Presidente e, per suo tramite, chiaramente le critiche sono rivolte a chi ha detto qualcosa di diverso. l'incremento dei fondi per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco. Questo incremento, che non è abbastanza sottolineato, rappresenta per noi anche l'occasione per ringraziare,

il collega Garavaglia, noi oggi abbiamo a disposizione, per quanto riguarda il 2025, soltanto 30 miliardi per poter gestire, come manovra libera, il bilancio e quindi la manovra finanziaria 2025; 30 2025, 35 nel 2026 e 40 nel 2027. Questo a causa dei tagli sul bilancio dovuti alla rata che dobbiamo pagare a causa del superbonus male applicato da parte vostra, altrimenti ci sarebbe stato il doppio

proprio perché abbiamo una visione dello Stato e dei cittadini diversa dalla vostra, più della metà, 15 miliardi, sono utilizzati per il taglio del cuneo fiscale e per il mantenimento delle tre aliquote aliquote Irpef. Noi continuiamo ad abbattere il cuneo fiscale e quindi a rendere strutturale una manovra anche culturalmente educativa rispetto a quella di regalare denari, soldi ed economia a chi sta seduto su un divano. È una visione diversa dello Stato e dei cittadini e in particolar modo diversa rispetto a quello che noi desideriamo sia il futuro dei nostri giovani. Ci saranno poi

dimostrare con i fatti un taglio sulla sanità. C'è stato anche un osservatorio della università Cattolica di qualche giorno fa che documenta un sensibile aumento rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti. Quando nel 2024 ci sono 134 miliardi, nel 2025 ci sono 136,5 miliardi e 140 miliardi nel 2026, significa che noi non abbiamo ridotto, bensì aumentato lo stanziamento sul Fondo sanitario nazionale. Dentro le tasche degli degli italiani ci sono più soldi: dai 1.900 euro *pro capite* a disposizione dei cittadini arriviamo a 2.300 euro *pro capite*. *(Applausi)*. Questi sono i fondi. Sempre per andare a citare quella famosa canzone di De Andrè, che diceva che

sono stati certificati 37 miliardi di tagli sulla sanità, e non mi risulta che dal 2010 al 2019 ci fosse il Governo di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e del centrodestra.

quella. Siamo i primi in Europa nell'applicazione del PNRR. Il fatto che siamo i primi a ricevere la sesta rata del PNRR dimostra la nostra capacità di saper fare politica e di saper fare risultato in Italia e nel mondo. Noi siamo quelli del *record* dell'occupazione, siamo quelli del *record* nella lotta all'evasione fiscale, siamo quelli elogiati dalla Commissione europea, siamo quelli che tengono la barra dritta nonostante il cambio della contabilità in Europa ci metta in difficoltà. *(Applausi)*. Noi abbiamo oggi il vice presidente Fitto che farà una battaglia per cambiare regole che penalizzano la nostra Nazione; regole mai cambiate da Governi che sono stati sempre troppo disposti e disponibili rispetto a regole che scrivevano i grandi dell'Europa, la Francia e la Germania. Noi non accettiamo che siano quelli i grandi, non accettiamo che siano la Francia e la Germania a scrivere le regole e ci candidiamo ad essere noi a scrivere le vere regole. Siamo quelli che registrano l'innalzamento del PIL rispetto alle altre Nazioni europee. Ricordo, ancora, il rialzo degli indici della borsa, l'abbassamento dello *spread*, il *record* di richiesta dei titoli di Stato. Moody's dice che stiamo sfiorando l'1 per Ho sentito dire in quest'Aula che Fitto sarebbe stato un'operazione sbagliata della Meloni, perché oggi Raffaele Fitto è esiliato in Europa. Raffaele Fitto è la vittoria strategica politica più intelligente del presidente Meloni, su cui nessuno di voi credeva o aveva scommesso. Già avevate preparato cartelli e comunicati stampa per andare a criticare un'operazione sbagliata da Giorgia Meloni in Europa. Anche in questo caso i gufi sono stati smentiti e oggi si stanno leccando le ferite.

ma l'analfabetismo non è soltanto fiscale, ma anche politico, economico e strategico su quella che è l'Italia e su quella che è la visione dell'Italia, che oggi si candida - ripeto - ad essere un interlocutore credibile in Europa e nel mondo. Noi siamo coscienti di non piacere al centrosinistra, di non piacere alla CGIL e di non piacere a Landini; siamo orgogliosi di non piacere a voi e siamo orgogliosi di piacere ai cittadini italiani, gli unici nostri giudici

di una chiara visione politica; tutti oggi sanno qual è la visione politica della *premier* Giorgia Meloni, mentre nessuno conosceva prima la visione politica dello Stato italiano, del Governo italiano, della Nazione Italia. Noi siamo quelli a protezione del ceto medio e degli indigenti. Noi siamo quelli - e ringrazio tutta la Commissione che hanno immaginato una nuova distribuzione del *payback* a favore delle Regioni più penalizzate dalla vecchia spartizione. Noi siamo quelli che oggi

con un'azione parlamentare di interlocuzione, il provvedimento in esame. Noi continuiamo a parlare e a piacere agli italiani, mentre voi continuate a parlarvi addosso e non vi capisce più nessuno. Fratelli d'Italia è a favore di questo provvedimento e ringrazia il Governo Meloni, ringrazia Giorgia Meloni, ringrazia il centrodestra. Andiamo avanti così, più convinti di prima.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Spinelli.

una grottesca, inopinata, minacciosa lezione di giornalismo a chi è stato accusato di spargere veleno, di fare dei piccoli pettegolezzi e di superficialità, con tanto di assai poco istituzionale gioia per il fatto che, a detta del Presidente, il giornale perderebbe copie su copie. Credo che i giornalisti del quotidiano «la Repubblica» non abbiano bisogno del fervorino e della mala pasqua di Rocca, sanno fare bene il proprio lavoro e certo non si lasceranno intimidire da chi usa indebitamente il proprio temporaneo potere per dare non richieste lezioncine di giornalismo. insultando «la Repubblica», Presidente, a un certo punto il presidente del Lazio la apostrofa come un giornale di *gossip*, come - e cito - «Cronaca vera», «Oggi» e «Gente». Solidarietà anche ai giornalisti di queste testate messi in un improbabile e surreale calderone da Rocca. Presidente, una libera vita democratica respira di tante cose, di senso delle istituzioni, che in questo caso è venuto meno, di autonomia e indipendenza dei media che al Governo e ai Governi, a chi è al potere, non solo possono, ma debbono essere sgraditi; i contropoteri di un ossigeno, insomma di un contesto che, giorno dopo giorno, strappo dopo strappo, abuso dopo abuso, rischia di far morire di asfissia e di malaria la nostra democrazia. Attenzione. Signor Presidente, è notizia di qualche ora fa che la corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, pronunciandosi sull'appello-*bis* sul femminicidio di Lorena Quaranta, ha confermato la condanna all'ergastolo per il suo assassino. È una notizia che rende il senso della giustizia e dimostra che la fiducia nella giustizia non è mai mal riposta. Il rischio elevatissimo era che si facesse strada un orientamento per il quale potevano entrare nei giudizi per femminicidio le valutazioni e il riconoscimento di attenuanti generiche. In questo caso la richiesta era l'attenuante generica per lo stress da contagio Covid; domani avrebbe potuto essere lo stress perché l'imputato era stato licenziato, perché aveva una doppia vita o temeva di essere scoperto. di un rischio elevatissimo, sul quale avevo sollecitato l'attenzione da parte del ministro Nordio presentando un'interrogazione, alla quale il Ministro ha risposto a ottobre, condividendo i miei stessi timori, informandosi specificatamente sulla vicenda giudiziaria, acquisendo una relazione, ma soprattutto dandomi conferma che saranno presto sviluppate delle linee guida per la formazione dei magistrati chiamati a pronunciarsi proprio nei processi per le violenze sulle donne, al fine di scongiurare il rischio che al danno già sofferto dalla vittima se ne aggiunga uno ulteriore di vittimizzazione secondaria. Esprimo quindi grande soddisfazione per la sentenza. Si chiude una pagina dolorosissima dal punto di vista giudiziario. Si chiude la vicenda giudiziaria, resta ovviamente la sofferenza umana della famiglia e dei genitori di Lorena Quaranta. Per tutte le donne che sono e continuano a essere, purtroppo, vittime di questa odiosa forma di violenza, contro la quale noi, come legislatori, dobbiamo continuare a impegnarci, ringrazio nuovamente e formalmente il ministro Nordio per l'attenzione e la sensibilità che ha dimostrato sul tema. Sono convinta che questa sentenza, che arriva a pochi giorni dal 25 novembre, subito dopo quella che c'è stata ieri nel processo contro Impagnatiello, sia un senso elevato della giustizia con la g maiuscola.